Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 28 gennaio 2010. Il ministro Alfano svolgerà ora la Relazione sull'amministrazione della giustizia. Subito dopo il suo intervento la seduta sarà sospesa per un'ora per consentire ai Gruppi un'approfondita valutazione delle sue comunicazioni. Entro la fine della discussione generale, per la quale sono state ripartite tre ore, dovranno essere presentate le proposte di risoluzione. Le dichiarazioni di voto e il voto degli strumenti di indirizzo avranno luogo entro questa sera, presumibilmente in un orario compreso tra le ore 21 e le ore 22. All'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani saranno posti disegni di legge di ratifica di accordi internazionali, tra cui quella concernente gli animali da compagnia, nonché il disegno di legge sulle cure palliative, ove concluso dalla Commissione. La prossima settimana, a partire dal pomeriggio di martedì 26 gennaio, il calendario prevede, oltre all'eventuale seguito del disegno di legge sulle cure palliative, la discussione della legge comunitaria, per la quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 6, del Regolamento. giornata di martedì 26 gennaio sarà nuovamente convocata la Conferenza dei Capigruppo al fine di definire la calendarizzazione, nella settimana compresa tra il 2 e il 4 febbraio, dei decreti-legge in scadenza in materia ambientale e proroga termini, nonché di valutare, alla luce dell'andamento dei lavori, l'integrazione del calendario della prossima settimana o di quella successiva con la discussione di mozioni sollecitate dai Gruppi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche quest'anno ho l'alto onore di riferire in quest'Aula sull'attività del Dicastero che rappresento e del Governo in materia di giustizia e di evidenziare i provvedimenti adottati in attuazione dell'indirizzo politico approvato dalla maggioranza degli italiani che ci hanno affidato la responsabilità di governare il Paese. Prima di tutto, desidero rivolgere un ringraziamento al signor Presidente della Repubblica, Capo dello Stato, Presidente del Consiglio superiore della magistratura e garante dell'unità nazionale, per la saggezza che ha avuto modo di dimostrare intervenendo nella delicata materia della giustizia, pronunziando parole sempre decisive per il mantenimento dei necessari equilibri istituzionali. Lo scorso anno ero partito dalla individuazione del più insidioso dei nemici della giustizia: l'insopportabile lentezza nell'affermazione giudiziaria delle ragioni e dei torti, della innocenza o della colpevolezza, che ha fatto del nostro Paese un luogo in cui la durata eccessiva dei processi disincentiva financo gli investimenti stranieri. Tutto questo accade malgrado diverse migliaia di magistrati, avvocati e personale giudiziario fanno quanto è nelle loro possibilità per adempiere al proprio dovere. Oggi sono qui per dire che la lentezza è nemico insidioso ma che si può vincere e il Governo ha la strategia per riuscirvi. Alcuni dati fotografano lo stato della giustizia in Italia, le cifre chiave della giustizia in Italia. 5.625.057 sono i procedimenti civili pendenti, con un aumento del 3 per cento rispetto al 2008; 3.270.979 quelli penali, con una riduzione modesta rispetto all'anno precedente; 65.067 detenuti (di cui 24.152 stranieri) si trovano reclusi nelle 204 strutture penitenziarie del nostro Paese; 20.959 minorenni sono segnalati dall'autorità giudiziaria minorile agli uffici di servizio sociale per i minorenni, con una crescente incidenza dei fenomeni di devianza minorile straniera. Questa enorme mole di lavoro - che non ha eguali negli altri Paesi dell'Unione europea - viene gestita da 9.080 magistrati togati (6.402 giudici e 2.090 pubblici ministeri); 3.513 giudici onorari; 40.456 unità di personale giudiziario; 1.399 addetti al settore minorile; 46.662 dipendenti dell'amministrazione penitenziaria. ben 5.183 (circa il 12 per cento) sono impegnati ad effettuare 28 milioni di notifiche manuali ogni anno (pari a 112.000 notifiche al giorno), di cui oltre la metà destinate agli avvocati. Circa il 12 per cento dei soli processi penali viene rinviato per omessa o irregolare notifica e lo stesso processo penale brucia, in media, 80 milioni di euro ogni anno per dichiarare prescritti 170.000 processi (cioè 465 al giorno, festivi compresi). Oltre 30.000 cittadini hanno chiesto di essere indennizzati a causa dell'irragionevole durata del processo, ottenendo decine di milioni di euro di risarcimenti, con un *trend* di crescita delle richieste pari al 40 per La giustizia costa 8 miliardi di euro l'anno, cioè circa 30 milioni di euro per ogni giornata lavorativa. La giustizia italiana è, dunque, in crisi. Per esprimere questo giudizio e formulare questa diagnosi non era necessario pronunziare questa relazione oggi. Sono qui a dirvi, dunque, non solo la diagnosi, ma la nostra terapia. In questo quadro, l'azione che ho avviato rispetta tre linee guida essenziali: l'adozione di misure organizzative; innovazioni legislative in materia sia ordinamentale che procedurale; previsione di un programma di impegni per l'anno 2010. Ed in tal senso proseguirò nella mia relazione illustrando, anzitutto, per ogni singolo settore, gli interventi svolti e i risultati ottenuti. Ma prima di ogni cosa desidero evidenziare gli straordinari risultati conseguiti dal Ministero della giustizia all'Aquila, in esito al tragico terremoto del 6 aprile 2009, poiché per la prima volta in epoca repubblicana (l'unico precedente risale, infatti, al terremoto di Messina del 1908) si sono resi contemporaneamente inutilizzabili tutti gli uffici giudiziari del distretto, insieme alla modernissima sala *server*, inaugurata pochi mesi prima del sisma, dove erano allocati dati essenziali e riservati. Ebbene, con uno sforzo eccezionale, dopo due giorni si è organizzato un efficiente servizio provvisorio per gli affari urgenti ed in soli 47 giorni si è messa in opera una nuova sede (in località Bazzano), interamente cablata ed informatizzata. Si è così restituito il servizio giustizia a una intera Regione, garantendo la trattazione dei procedimenti in grado di appello relativi agli altri tribunali del distretto. Rivendico con soddisfazione ed emozione questo tributo dovuto ai tanti aquilani che hanno perso affetti, lavoro e proprietà, e sono fiero di aver preteso ed ottenuto che gli uffici giudiziari riprendessero a funzionare proprio all'Aquila. Il mio impegno non si è esaurito qui, poiché nei prossimi 24 mesi restituiremo alla funzione giudiziaria il palazzo di giustizia gravemente danneggiato e sarò, inoltre, personalmente presente, avendo scelto quella sede, all'Aquila, il 30 gennaio prossimo, alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario. La prima parte di questa Relazione vuole riferire all'Aula le misure di efficienza che il Governo ha adottato in quest'anno per far funzionare meglio il servizio giustizia. Abbiamo

Avevo già affermato, lo scorso anno, che il Ministro della giustizia deve riappropriarsi della funzione organizzativa che l'articolo 110 della Costituzione gli affida e dissi che l'autonomia e l'indipendenza dei giudici non può scindersi dall'efficienza del servizio, precisando che non può chiedersi al Ministro di essere responsabile del servizio giustizia senza che lo stesso Ministro abbia potestà organizzative effettive. Ebbene, questo percorso nello scorso anno ha avuto un forte e positivo impulso pervenendo a risultati significativi. Come primo aspetto, vorrei parlare del piano nazionale di diffusione delle cosiddette *best practices*. Sul piano amministrativo, il piano nazionale di diffusione di queste migliori pratiche coinvolge ormai circa un centinaio di uffici giudiziari. È stato definito il progetto di «Diffusione del modello di autoanalisi e miglioramento del servizio giustizia», realizzandosi una versione personalizzata per il sistema giudiziario. Sarà possibile ora attenuare le differenze di rendimento che danno luogo ad una giustizia che si muove a macchia di leopardo, con una inaccettabile disarmonia di trattamento dei cittadini destinatari di un servizio che, a seconda della sede, dà risposte differenti e che, a legislazione invariata - essendo le leggi tutte uguali da Lampedusa a Trento - e a parità di risorse e magari a parità di problemi, fornisce ottimi livelli di efficienza ovvero ritardi e disservizi inaccettabili. Le differenze possono essere clamorose, come in due tribunali del Nord-Italia distanti solo 70 chilometri, dove il primo raggiunge un indice di smaltimento di smaltimento dell'arretrato del 148 per cento, dimezzando la pendenza dell'ultimo quinquennio, mentre il secondo, nello stesso periodo, vede esplodere il numero dei procedimenti arretrati. Tali divergenze dipendono da *deficit* di tipo organizzativo e, talvolta, da una scarsa capacità manageriale e di *leadership* del capo dell'ufficio. Oggi la temporaneità degli incarichi direttivi e la verifica richiesta dalla legge dopo il primo quadriennio di dirigenza offre una importante opportunità al CSM per una efficace selezione dei capi degli uffici, che si spera non condizionata da logiche correntizie e corporative. In questa logica, proponiamo una nuova cultura della dirigenza negli uffici giudiziari. Ed è questo il secondo aspetto. Per il recupero dell'efficienza del sistema occorrono interventi radicali anche sul piano legislativo e ordinamentale, finalizzati ad affermare il primato della professionalità gestionale e organizzativa dei dirigenti degli uffici. Pende in Commissione giustizia, proprio qui al Senato, il disegno di legge n. 1440, di iniziativa governativa, che contiene norme che esprimono una nuova cultura della dirigenza negli uffici di giudiziari. È ben noto che un ottimo magistrato può rivelarsi un pessimo dirigente. Per questo abbiamo previsto una formazione specifica per i magistrati che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi, con corsi mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse, e abbiamo previsto l'obbligo per il magistrato dirigente di vigilare sul rispetto dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero. Si è poi previsto che il concerto espresso al CSM dal Ministro per il conferimento degli incarichi direttivi deve essere motivato con riferimento alle capacità organizzative e che tale specifica valutazione sia estesa alla conferma delle funzioni di direzione degli uffici giudiziari dopo il primo quadriennio. Un terzo aspetto di natura organizzatoria lo inseriamo nell'ambito degli interventi in materia di costi e di disciplina delle intercettazioni. Due sono le questioni di particolare importanza che poniamo a base del nostro intervento: la garanzia della *privacy* dei cittadini, evitando degenerazioni, eccessi e abusi nell'uso di uno strumento particolarmente delicato ed invasivo; la necessità di razionalizzare i costi di un servizio che, sino allo scorso anno, era sostanzialmente fuori controllo. Nell'ottobre del 2008 ho constatato un debito contratto dal Ministero nei confronti di società che gestiscono i servizi di intercettazione a partire dal 2006 pari a quasi cinquecento milioni di euro. Gli amministratori di queste società minacciavano, in caso di ulteriore morosità, l'interruzione dei servizi, con intuibili conseguenze gravissime sulle indagini in corso. L'immediata azione del mio Dicastero non solo ha fatto sì che i debiti pregressi fossero onorati ma, attraverso l'istituzione di una unità di monitoraggio sulle spese per le intercettazioni, ha evidenziato come il Ministero pagasse, per medesime prestazioni, da 4 a 25 euro al giorno per ogni singola intercettazione telefonica. La presa d'atto di questo ingiustificabile spreco del denaro dei contribuenti e le verifiche disposte hanno determinato nel corso del 2009 un abbattimento della spesa, senza incidere sulla quantità di intercettazioni disposte, con un risparmio dei costi unitari erogati dall'amministrazione stimabile nell'ordine del 25-30 Si è poi proceduto anche alla creazione di un apposito capitolo di bilancio per sganciare le procedure di pagamento di queste spese dal capitolo generale. Oggi, dopo la larga approvazione presso la Camera dei deputati del disegno di legge di riforma del sistema delle intercettazioni, il Governo aspira ad una sua rapida e definitiva approvazione. La concentrazione delle operazioni di registrazione a livello distrettuale e la previsione di un termine di durata massima delle intercettazioni determineranno una ulteriore diminuzione dei costi ed una più responsabile ed attenta gestione di tale strumento investigativo. Quanto al merito delle scelte operate, desidero ribadire ancora una volta che il rafforzamento del sistema del cosiddetto doppio binario lascia inalterato l'utilizzo della strumento per i reati in materia di criminalità organizzata e terrorismo. Un quarto aspetto riguarda, in tema di efficienza, gli interventi in materia di cosiddette sedi disagiate. Prima di illustrare quanto fatto dal Governo Berlusconi per risolvere il problema delle sedi giudiziarie sgradite ai magistrati, appare necessario sgombrare il campo da una mistificazione. Non si tratta di un problema che nasce in questa legislatura, ma che affligge da sempre il sistema giudiziario. Le cause di questa situazione sono da ricondursi: al fatto che ci sono sedi che sistematicamente non vengono scelte dai magistrati; alla prassi del CSM di destinare tali sedi ai magistrati di prima nomina; alla conseguente fuga verso altri lidi, non appena possibile, degli stessi magistrati; alla rigidità del sistema di mobilità dei magistrati. In questo contesto, il divieto di destinazione dei magistrati di prima nomina all'esercizio di funzioni monocratiche - introdotto nella precedente legislatura da una diversa maggioranza - non ha determinato effetti catastrofici ma, semmai, possiede il merito di eliminare il cronico ed imperante nonnismo giudiziario. In pratica per decenni si è, da un lato, provveduto alla copertura delle sedi sgradite con gli ultimi arrivati e, dall'altro, dopo aver formato in tali sedi i giovani magistrati, si è loro garantita una sede più comoda proprio quando avrebbero potuto spendere efficacemente sul posto la professionalità acquisita. Il Governo è fattivamente intervenuto per porre rimedio a tale situazione e la migliore prova di ciò risiede nei due decreti-legge che, in poco più di un anno, sono stati dedicati alla soluzione di questo problema. Il primo, adottato poco dopo l'esordio di questa legislatura, prevede incentivi anche economici per la copertura delle sedi. La normativa si è rivelata molto utile - poiché circa la metà dei posti messi a disposizione sono stati coperti - ma non è stata risolutiva. È stato pertanto necessario, nelle scorse settimane, emanare un nuovo decreto-legge riguardante "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario". Questo decreto ha introdotto un sistema di maggiore cogenza, che ha scatenato talune polemiche, alcune delle quali strumentali e fuori luogo. Mi riferisco alle norme relative al trasferimento d'ufficio nelle sedi sgradite. Si tratta di una normativa transitoria che trova un limite temporale nella data del 31 dicembre 2014, poiché entro tale termine andrà a regime la modifica ordinamentale oggi in discussione alla Camera, idonea a risolvere in via definitiva il problema. Si è anche proceduto, in quel contesto di decreto, ad un aumento del numero delle sedi annualmente individuabili come disagiate da parte del Consiglio superiore della magistratura (estese ad ottanta) nonché dei magistrati ivi destinabili (aumentati a Colgo l'occasione per comunicare che, alla presenza del sottosegretario Caliendo qui presente, poc'anzi in Commissione giustizia alla Camera dei deputati è stato votato un emendamento proposto dalle forze di opposizione e riformulato dal Governo che ha trovato una larga convergenza. Pertanto,

Devo, inoltre, riferire - questo è un quinto argomento in materia di efficienza - gli interventi in materia di digitalizzazione del sistema giudiziario poiché il decreto-legge riguardante "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario", il medesimo col quale abbiamo affrontato la questione delle cosiddette sedi disagiate, contiene disposizioni per assicurare risparmi di spesa e l'abbattimento dei tempi del processo. Mi riferisco all'anticipazione dell'entrata in vigore del processo telematico che completa la digitalizzazione della giustizia, applicando l'informatica a tutti gli atti del processo, civile e penale. Lo abbiamo fatto con decreto-legge per far sì che entrasse immediatamente in vigore nell'ordinamento giuridico. In particolare, si rendono immediatamente applicabili le comunicazioni e le notificazioni telematiche tra uffici giudiziari e avvocati ed infatti, salvo che per le notifiche agli imputati, sarà possibile utilizzare sempre la posta elettronica certificata. Su questi interventi mi aspetto una larghissima condivisione di tutte le forze parlamentari trattandosi di innovazioni sostanzialmente condivise. L'obiettivo finale è quello di realizzare un'unica «piattaforma di servizi documentali» che consentirà una drastica riduzione del cartaceo, l'abbattimento dei costi e la velocizzazione di tutte le procedure. Lo scorso anno avevo anticipato - è questo il sesto argomento - che il recupero di efficienza e la razionalizzazione delle risorse disponibili passava anche dalla operatività del Fondo unico giustizia. Com'è noto, confluiscono nel fondo le somme di denaro e i proventi sequestrati, confiscati o depositati nell'ambito di procedimenti civili, penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione. Questo innovativo strumento assicura una pronta disponibilità delle risorse da reinvestire nel sistema giustizia, di cui ottimizza la gestione anche sotto il profilo finanziario. Ho il piacere di comunicare a quest'Aula che oggi sono già confluiti nel Fondo unico giustizia 1 miliardo e 590 milioni di euro somma nell'ambito della quale si evidenziano 631,4 milioni di euro disponibili per la riassegnazione *pro quota* al settore giustizia. Ben può dirsi, dunque, che anche questa è una scommessa vinta, grazie a un complesso e intenso lavoro del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, della Presidenza del Consiglio, che ha condotto all'emanazione del regolamento con decreto interministeriale del luglio 2009. Un ultimo aspetto in questa parte riguarda la gestione del personale amministrativo. Il 16 dicembre, dopo dieci anni di attesa, è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo

Si tratta di una prima fondamentale tappa per il raggiungimento dell'obiettivo dell'efficienza della macchina giudiziaria perseguito anche attraverso la valorizzazione del personale dell'amministrazione giudiziaria. Molto rimane ancora da fare per l'adeguamento degli organici, per la ottimale distribuzione sul territorio nazionale, per implementare ulteriormente le procedure di valorizzazione e per il riconoscimento sia economico che giuridico delle professionalità acquisite. Proprio per queste ragioni, sento la necessità di ribadire, in questa solenne occasione e nel luogo in cui risiede la sovranità popolare, il mio sentito ringraziamento a tutti i dirigenti e a tutto il personale amministrativo, che continua a dare quotidiana prova di grande professionalità e di spirito di servizio. Esaurita la parte che riguarda l'efficienza del sistema giustizia e i sette pilastri su cui abbiamo fatto la scelta di poggiare la nuova efficienza del sistema giustizia (pilastri non tutti edificati per intero, ma la cui edificazione è già certamente avviata), vorrei dedicarmi alle alle attività legislative che si sono svolte. Infatti, tornando a distanza di un anno in un'Aula parlamentare, ho il dovere di riferire ciò che ha

sia sul piano bilaterale che su quello della partecipazione agli organismi internazionali, dove sempre di più si forma il diritto in Europa. Il 2009 è stato contrassegnato in primo luogo dalla Presidenza italiana del G8, G8, evento di rilevanza mondiale sui temi della lotta alla criminalità organizzata e sulle strategie internazionali nella lotta al terrorismo. L'obiettivo finale di una strategia unitaria da parte della comunità internazionale è stato raggiunto nella Conferenza ministeriale dei Ministri della giustizia e degli affari interni che ha avuto luogo a Roma il 29 e 30 maggio scorso, il cui più importante risultato è stata la dichiarazione finale, sottoscritta da tutti i Ministri, da tutti i Ministri, che ha adottato il modello di legislazione italiana in materia di aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati come rotta e modello di riferimento. Particolarmente rilevante è stata, poi, la partecipazione alle attività dell'Unione europea nel settore della giustizia e degli affari interni e cioè al Consiglio di giustizia e degli affari interni (il Consiglio GAI), così com'è costantemente fattiva la collaborazione al programma di Stoccolma: nel 2009 abbiamo svolto sei Consigli GAI e venti incontri bilaterali, in Italia ed all'estero, oltre a due vertici bilaterali e a due conferenze multilaterali. multilaterali. Ho avuto modo di incontrare vari Ministri: tra gli altri quelli del Canada e degli Stati Uniti, Governo quest'ultimo con cui si è affrontata la vicenda dei detenuti di Guantanamo, tre dei quali sono stati accolti nelle nostre strutture penitenziarie. Intensi anche i rapporti con il Ministero della giustizia russo, dai quali ha preso avvio una preziosa attività di cooperazione, culminata nel Vertice italo-russo tenutosi alla Farnesina nel dicembre Nel prossimo futuro - e, se possibile, in quest'anno 2010 - è mia intenzione trovare modi e forme per porre l'Italia al centro del dialogo tra gli ordinamenti giuridici dei Paesi del Mediterraneo per contribuire, attraverso tale dialogo, ad un nuovo percorso di pace nell'area. Passando ora ai provvedimenti legislativi, desidero ricordare che lo scorso anno avevo sottoposto alla vostra attenzione un elenco di settori su cui intervenire, per consentire allo Stato di fornire al cittadino utente del servizio giustizia una risposta certa, pronta ed efficace nel riconoscimento dei propri diritti. Avevo così distinto precise linee d'intervento riguardanti il processo civile, il processo penale, le norme antimafia, gli interventi sul sistema carcerario, la riforma della magistratura onoraria, la riforma delle professioni del comparto giuridico-economico. Questi erano gli impegni di un programma ambizioso, impegnativo e caratterizzato da un percorso attuativo denso di ostacoli e fonte di polemiche, ben al di là del legittimo del legittimo ed aspro confronto parlamentare tra le forze politiche della maggioranza e dell'opposizione. È un programma che, in massima parte, possiamo dire realizzato: e la parte che non è stata ancora realizzata è certamente già avviata. a cominciare dalla giustizia civile. Infatti, a fronte della intollerabile lentezza e farraginosità della giustizia civile, su iniziativa del Ministero della giustizia, nel giugno del 2009 è stata approvata dal Parlamento la legge 18 giugno 2009, n. 69 (la cosiddetta riforma del processo civile), ispirata al contenimento dei tempi del giudizio. In questo senso, è stata prevista una nuova disciplina delle spese processuali, per ridurre la litigiosità e sanzionare le parti che abusano del processo, cagionando danni sia alla controparte sia all'amministrazione giudiziaria. Per ridurre i tempi del processo è stata operata una diffusa riduzione dei termini collocati nel codice di procedura civile. È stato introdotto l'istituto del filtro in Cassazione, che limita l'acceso nei procedimenti al giudizio di legittimità ai soli casi necessari; nonché quello dell'*astreinte*, volto a disincentivare, con le penalità anche risarcitorie prefissate dal giudice, inadempimenti non facilmente sanzionabili quali quelli degli obblighi di fare infungibile o di non fare. Vorrei ricordare in quest'Aula che tale norma ha già trovato applicazione da parte dei giudici del nostro Paese. La stessa legge ha poi conferito delega al Governo per la disciplina di un ulteriore istituto fondamentale per la deflazione dei processi civili: la mediazione finalizzata alla conciliazione. La mediazione ha lo scopo di evitare la controversia, come già accade in altri Paesi ed in coerenza con una direttiva dell'Unione europea. La delega ha già trovato attuazione mediante l'approvazione del Consiglio dei ministri del relativo decreto e si attende il parere delle competenti Commissioni parlamentari per procedere alla sua approvazione definitiva. riguarda la materia penale, un'espressa citazione il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, che ha introdotto, tra i delitti contro la libertà morale, il nuovo reato di atti persecutori (il cosiddetto *stalking*),

In materia di sicurezza pubblica, la legge 15 luglio 2009, n. 94, è intervenuta per reprimere la particolare efferatezza e diffusione di alcuni fenomeni delinquenziali, nell'ottica della tutela della sicurezza dei cittadini. Le nuove norme - voglio ricordarlo - assicurano, tra l'altro, la difesa dei minori e dei disabili, prevedendo anche un rafforzamento del contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina. Tra le tante innovazioni, meritano una speciale citazione: l'aggravante per i delitti contro il patrimonio commessi in danno di soggetto portatore di minorazione fisica, psichica o sensoriale; l'aggravante per i soggetti adulti che commettono il reato in concorso con minorenni; il delitto di impiego di minori nell'accattonaggio; l'aggravante per il delitto di violenza sessuale commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di istituti d'istruzione o di formazione frequentati dalla persona offesa; l'innalzamento della pena per il delitto di violazione di domicilio; l'arresto obbligatorio nei casi di furto commesso da soggetto che porta indosso armi o narcotici, senza farne uso, ovvero da tre o più persone; l'introduzione della truffa aggravata ai danni di soggetti deboli o anziani. Sono

Nel contrasto alla criminalità di stampo mafioso, il Governo Berlusconi ha varato, nei primi 20 mesi, il più efficace e rilevante pacchetto di norme antimafia dai tempi successivi alle stragi di Capaci e di via D'Amelio. 2009, n. 94, il cosiddetto pacchetto sicurezza, contiene importanti modifiche in materia sostanziale, in materia di misure di prevenzione antimafia, di sequestro e confisca, così come nella materia dell'ordinamento penitenziario. Tale legge introduce due nuove figure di reato volte ad arricchire la punibilità delle condotte rilevanti nel sostegno illecito delle associazioni mafiose, tra cui spicca il nuovo articolo 391-*bis* del codice penale, che punisce l'attività di chiunque consente a un detenuto sottoposto a particolari restrizioni di comunicare con altri. Ma, soprattutto, la legge n. 94 del 2009 fornisce alle forze dell'ordine ed alla magistratura strumenti di straordinaria efficacia nell'azione di recupero dei beni frutto delle attività criminali delle associazioni mafiose, ampliando l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione. Si prevede che le misure di sicurezza patrimoniali possono essere applicate indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto: il principio è che, se si deve colpire il bene in quanto pericoloso in sé, lo si può fare al di là della pericolosità del soggetto cui quel bene appartiene. In tema di sequestro e confisca, si è proceduto al rafforzamento delle ipotesi di cosiddetta confisca estesa, di modo che - disperso il denaro o i beni illecitamente acquisiti - il giudice può ordinare la confisca per un valore equivalente, incidendo sul patrimonio posseduto dal reo anche per interposta persona. Vengono finalmente disciplinate in modo chiaro le modalità di esecuzione dei sequestri preventivi e viene istituito l'albo nazionale degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati, che garantirà una specifica professionalità nella gestione dei beni sottratti alla criminalità organizzata in grado, dunque, di produrre economie legali, assicurando il mantenimento dei posti di lavoro. Le Forze di polizia saranno dotate dei beni mobili registrati sequestrati che potranno essere loro affidati per lo svolgimento dei compiti di istituto. Molto importanti sono anche le altre misure di natura amministrativa, introdotte con la legge sulla sicurezza pubblica. Al fine di prevenire le infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, è attribuito al prefetto il potere di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri. Infine, la legge modifica la normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali a causa di infiltrazioni e di condizionamenti di tipo mafioso. Queste modifiche legislative stanno già producendo risultati straordinari, mai conseguiti in passato, dei quali le forze dell'ordine e la magistratura sono le prime testimoni e protagoniste. La imponente mole di sequestri e confische definitive operata anche in queste ultime settimane (e financo stamattina a Napoli) dimostra il concreto valore di questi provvedimenti e l'azione dello Stato sarà anzi rilanciata di fronte a tanto violente quanto vili forme di reazione. Ne è prova l'azione ferma, immediata ed efficace del Governo Berlusconi in risposta ai recenti e gravi fatti di Reggio Calabria. In tal senso, il mio Dicastero ha già avviato le procedure per incrementare gli organici degli uffici giudiziari di Reggio Calabria, dotandoli di due posti in più sia nella procura generale che nella procura della Repubblica e nel tribunale. In conclusione di questo capitolo riguardante le norme antimafia, in questa circostanza e in questa occasione voglio dare atto al Senato della Repubblica e a tutte le forze politiche qui presenti di avere contribuito (maggioranza e opposizione insieme) all'irrobustimento del disegno del Governo, così come era venuto fuori dal Consiglio dei Ministri, essendo stato il passaggio al Senato un passaggio fortemente virtuoso che ha consentito alla legge di diventare efficace così come ho tentato di rappresentarla. Veniamo ora al sistema carcerario. La situazione carceraria nel nostro Paese mi ha spinto, il 13 gennaio scorso, a chiedere la dichiarazione da parte del Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza fino a tutto il 2010. Svanito l'illusorio effetto dell'indulto del 2006 in conseguenza del *trend* continuamente crescente degli ingressi nelle carceri del nostro Paese, la dichiarazione dello stato di emergenza costituisce uno strumento fondamentale per provvedere ad interventi strutturali di medio e lungo periodo, che consentano di rispettare il precetto dell'articolo 27 della Costituzione, che - vorrei ricordarlo - prevede che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Il Piano carceri che scaturirà dagli atti conseguenti alla dichiarazione di emergenza si poggia su altri tre pilastri fondamentali: gli interventi di edilizia penitenziaria per la costruzione, in prima battuta, di 47 nuovi padiglioni

delle persone imputabili per reati fino a tre anni, che potranno così svolgere lavori di pubblica utilità; l'assunzione di 2.000 nuovi agenti di polizia penitenziaria. A partire dal 2011, poi, saranno realizzate le altre strutture previste dal Piano. Complessivamente, tali interventi porteranno alla creazione di 21.709 nuovi posti negli istituti penitenziari e al raggiungimento di una capienza totale di 80.000 unità. Per realizzare tutto ciò, saranno utilizzati 500 milioni di euro già stanziati in finanziaria e altri 100 milioni di euro provenienti dal bilancio della giustizia. Parallelamente a questo intervento, ho avviato, con l'appoggio del Vice Presidente della Commissione europea, del Ministro della giustizia spagnolo e del Ministro della giustizia svedese (gli ultimi due Paesi che hanno ricoperto il semestre di presidenza europeo), un'azione europea per dare soluzioni concrete a quei Paesi nei quali il problema del sovraffollamento nelle carceri è determinato anche dalla massiccia presenza di detenuti stranieri. Il mio obiettivo è quello di ottenere il trasferimento dei detenuti nei loro Paesi d'origine e di giungere all'elaborazione di un Piano europeo per le carceri, anche tramite fondi dell'Unione. Nel quadro Nel quadro dell'approvazione del «Programma di Stoccolma 2010-2014 per un'area europea di libertà, di sicurezza e giustizia», il Parlamento europeo ha approvato nel novembre scorso una risoluzione che getta le basi per il raggiungimento di tale duplice obiettivo. Questo è un risultato che porta l'*imprinting* del Governo italiano e del quale siamo fortemente soddisfatti. Il regime di cui all'articolo 41-*bis*, nell'ambito del sistema carcerario, riguarda oggi un totale di 645 detenuti. Le donne sottoposte a tale regime sono 3. Al 14 dicembre 2009, erano stati emessi 112 decreti ministeriali di prima applicazione, a fronte degli 87 emessi nel corso di tutto il 2008. Nell'ultimo anno il regime del carcere duro ha potuto trarre un notevole rafforzamento anche dalle novità introdotte dalla recente legge n. 94 del 2009. Si è infatti resa ancora più impermeabile la possibilità di contatto tra il mafioso detenuto e gli associati in libertà, allo scopo di stroncare ogni possibile forma di comunicazione sia interna che esterna. Inoltre, è stata introdotta una sostanziale innovazione dell'istituto, i cui punti più rilevanti sono: l'estensione della durata del provvedimento ministeriale e delle successive proroghe; la precisazione dei criteri cui il giudice si deve attenere nel valutare se disporre o meno la proroga stessa; l'accentramento della competenza in materia di reclamo in capo al tribunale di sorveglianza di Roma, per il quale è stata opportunamente avviata la procedura di aumento dell'organico. A riprova della funzione strategica ho inteso attribuire al regime detentivo speciale dell'articolo 41-*bis*, vi segnalo che - qualche giorno fa - in perfetta sincronia con la direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta ho disposto, nei confronti di cinque pericolosi esponenti della mafia nissena già detenuti, l'immediata applicazione del regime speciale, così contribuendo a sventare il progetto di attentato, ordito dagli stessi, contro un magistrato operante nella medesima sede giudiziaria. Ancora una volta, dunque, la collaborazione tra procura antimafia ed uffici ministeriali ha consentito di dare una risposta immediata nel contrasto alla mafia, dando prova dell'importanza dell'impegno unitario dello Stato contro la criminalità organizzata.

Noi intendiamo proporre innanzitutto un piano straordinario di smaltimento dell'arretrato civile; vogliamo dare una soluzione definitiva al problema dei vuoti di organico nelle sedi sgradite ai magistrati; inoltre: la riforma della magistratura onoraria; la riforma dell'avvocatura; la legge sulle intercettazioni; la riforma del processo penale; la riforma contemplata dal disegno di legge stamane approvato sulla ragionevole durata del processo penale, il quale, benché di iniziativa parlamentare, è sostenuto dal Governo in quanto, deflazionando il processo penale, produrrà ulteriori risparmi di spesa conseguenti all'azzeramento del rischio della legge Pinto, i cui costi come ho accennato in premessa - gravano in maniera pesante sul bilancio della giustizia a causa dell'indennizzo dovuto anche per la lunghezza del processo. intendiamo rispettare minuziosamente i termini delle altre deleghe che il Parlamento ha concesso al Governo in ambito di riforma del processo civile, tra le quali quelle per la semplificazione dei riti e la previsione dell'atto pubblico informatico. Così come da programma di Governo, intendiamo proporre al Parlamento il tribunale della famiglia, nonché un disegno di legge che renda migliore la legge sulle adozioni internazionali; vogliamo introdurre nel codice civile il contratto di fiducia e il contratto informatico; intendiamo attuare il principio di sussidiarietà mediante un'organica riforma degli enti giuridici di cui al libro I del codice civile.

legislativo. Per ultimo, ma non da ultimo, intendiamo proporre le riforme costituzionali della giustizia. Alcuni di questi argomenti meritano qualche approfondimento prima di rassegnare le mie conclusioni. il piano straordinario di smaltimento dell'arretrato civile, soltanto con l'alleggerimento dell'enorme fardello dei procedimenti arretrati sarà possibile ottenere concreti benefici dalla riforma del processo civile e dalle misure di efficienza che abbiamo portato avanti. L'analisi dei flussi consente di affermare che quei procedimenti che il sistema processuale si trova a gestire nascono nella Il sistema processuale riesce a smaltire quasi per intero il totale dei processi annualmente sopravvenuti: nel 2008, su 4.826.373 procedimenti sopravvenuti, quelli esauriti sono stati ben 4.605.551, con un saldo negativo di circa 220.000 processi (il 3 per cento di cui parlavo prima). Pertanto, vi è una quasi totale capacità del sistema giudiziario di smaltire sul piano quantitativo il numero dei processi civili che entrano nell'ambito di un anno solare. Il vero problema da risolvere è, quindi, quello dell'eliminazione dell'arretrato. Per questo motivo, presenterò in tempi brevi al Consiglio dei ministri il piano straordinario per lo smaltimento dell'arretrato civile. Anche quest'anno il rapporto *Doing Business* 2010, recentemente pubblicato dalla Banca mondiale, che vede l'Italia al 78° posto su 183 Nazioni, dimostra l'incidenza negativa del sistema giudiziario sugli investimenti di imprese straniere, mentre il *ranking* in materia di *enforcing contracts*, ossia dei contratti, vede precipitare l'Italia al 156° posto. Ecco perché abbiamo la consapevolezza e il dovere di considerare lo stato della giustizia civile una vera e propria emergenza nazionale, da affrontare con strumenti straordinari e fortemente innovativi, che proporrò al Consiglio dei ministri e in riferimento ai quali verrò a chiedere nuovamente il consenso del Parlamento. dai Gruppi* *PdL e LNP).* Sul fronte della magistratura onoraria, il Consiglio dei ministri è in procinto di varare un provvedimento di riordino complessivo del suo ruolo e delle sue funzioni, così come previsti dalla legge n. 127 del 2008, il cui esame è stato già avviato prima della sospensione natalizia. Il disegno di legge persegue l'obiettivo di attuare una riforma organica della magistratura onoraria, muovendosi lungo tre direttrici fondamentali: la predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari; la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari di tribunale; la riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace. L'intervento è altresì finalizzato a contenere la durata del processo entro il termine di ragionevole durata imposto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, attraverso una migliore organizzazione e gestione delle risorse disponibili. Puntiamo molto anche - presidente Berselli - sulla riforma delle professioni. Già lo scorso anno avevo riferito che il Governo aveva intenzione di procedere ad un'organica riforma delle professioni, coinvolgendo direttamente gli ordini degli avvocati, dei notai e dei commercialisti. Il confronto è iniziato da tempo ed è già stato elaborato un testo condiviso, che il Governo non ha voluto fare suo e presentarlo in Consiglio dei ministri al fine di lasciarlo al libero dibattito parlamentare, pur sostenendolo pienamente. Alcuni aspetti di tale Alcuni aspetti di tale disegno sono fortemente innovativi e danno luogo a nuove importanti garanzie per i cittadini utenti, come la disciplina delle società tra avvocati, e tra avvocati ed altri professionisti; la riserva esclusiva agli avvocati della difesa in ogni giudizio; il mantenimento dell'iscrizione all'albo condizionato dalla prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione; l'eliminazione dell'iscrizione automatica all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, condizionata ora al superamento di un esame o di un corso-concorso. Come si vede, è una riforma incentrata sulla qualità professionale ulteriormente rafforzata da nuove modalità di accesso alla professione. che ho illustrato offre, in conclusione, il senso di un'azione organica del Governo finalizzata a concretizzare un solenne impegno preso non soltanto con i nostri elettori ma con tutto il Paese: riformare un sistema giudiziario da troppo tempo malato ed autoreferenziale. Il tempo trascorso in questa prima parte di legislatura è servito a convincermi, definitivamente, che per ottenere risultati duraturi non basta un'azione di tipo ordinario, anche se attenta e scrupolosa. Occorre procedere alla riscrittura di alcune fondamentali e strategiche regole costituzionali che, ferma l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, attribuiscano al giudice il ruolo centrale nell'esercizio della giurisdizione e garantiscano ad un separato ordine dell'accusa piena autonomia nell'esercizio dell'azione penale nonché nello svolgimento delle indagini sulle notizie di reato che ad esso pervengano. Bisognerà, inoltre, prevedere le giuste procedure che consentano - fuori da ogni logica punitiva ma nello stesso tempo lontani da difese corporative - di affermare il binomio potere - responsabilità anche nell'esercizio della giurisdizione. In quest'ambito dovranno anche essere adeguate e ripensate la struttura, la composizione e la funzione del Consiglio superiore della magistratura, ben oltre l'esigenza di innovarne il sistema elettorale che, com'è noto, può essere modificato con legge ordinaria. Occorre, infatti, restituire, in concreto, al Consiglio superiore la sua funzione di organo di garanzia superando ogni equivoco su una malintesa sua funzione rappresentativa che non pare coerente neppure con il disegno originario dei nostri Padri costituenti e che, invece, si è insinuata troppo spesso nella prassi consiliare. Occorre, infine, garantire assoluta autonomia, separatezza ed esclusiva natura giurisdizionale anche riguardo alla sua composizione - alla giustizia disciplinare in modo da evitare le negative conseguenze di una giurisdizione domestica. Ed è con questi intendimenti che, onorevoli senatori, sono certo che, con il sostegno dei partiti e dei singoli parlamentari sensibili a questi temi, il 2010 possa passare alla storia come l'anno della compiuta come l'anno della compiuta riforma ordinaria e costituzionale del sistema giudiziario italiano. *(Applausi

signor Ministro, il Gruppo del PD presenterà una proposta di risoluzione per esprimere la propria insoddisfazione sulle comunicazioni che lei ha presentato poiché non dimostrano una visione strategica per risolvere i problemi della giustizia Non vi è dubbio che numerose siano le innovazioni apportate o messe in campo in materia di giustizia e sicurezza ma, oltre a non riflettere un progetto organico, non tutte sono davvero utili al bene comune e soprattutto rispettose di regole che, per anni, sono state considerate patrimonio irrinunciabile del Paese e riflettono i valori della nostra Costituzione. Tanto più che è sconfortante pensare che ai guasti potrà porre rimedio solo la Corte costituzionale, dopo, con le sue sentenze. Quella Corte il cui operato non viene politicamente accettato, ma criticato con pericolo per la democrazia nel Paese. Colpisce, poi, signor Ministro, che lei non abbia fatto alcun riferimento al contributo fornito dall'opposizione per la stesura di norme di contrasto alla criminalità organizzata, norme spesso estrapolate da testi o emendamenti predisposti da parlamentari del PD. Analogamente, nessun riconoscimento al contributo del PD alla legislazione di contrasto alla violenza alle donne, di fatto recepita dai nostri disegni di legge. Signor Ministro, il Governo di cui lei fa parte, nonostante da anni ne proclami la necessità, non ha ancora presentato un progetto organico di interventi. Il Governo continua, invece, ad insistere in logiche estemporanee ed emergenziali, caratterizzate in campo penale da un diritto securitario e da norme *ad personam*, così alimentando un contesto di permanente conflittualità, che tocca tempi e contenuti delle riforme a danno dei cittadini. In questo modo continuano a maturare le inefficienze del sistema e a manifestarsi aspri aspri contrasti fra politica e magistratura. Tutto ciò malgrado l'inefficienza della giustizia, testimoniata dall'impressionante numero dei procedimenti pendenti, influisca sul sistema economico e produttivo del Paese e richieda pertanto una linea strategica ben definita. Il protrarsi di una simile situazione di inerzia riformatrice (come tale definita dagli avvocati dell'Unione camere penali) non può essere ulteriormente tollerata né può essere consentito ricorrere, in luogo delle necessarie riforme, a provvedimenti «scorciatoia» quale il disegno di legge sul processo breve, oggi approvato dalla maggioranza al Senato.

nel giorno in cui in quest'Aula è stato approvato il processo breve, il signor Ministro della giustizia è venuto a rappresentarci un quadro dello stato della giustizia italiana fatto

ossia agli ultimi scandali finanziari e industriali, Bipop Carire, Opengate, Cirio, Parmalat, Lehman Brothers.

sono andati in prescrizione, cioè i banchieri che avevano frodato la buona fede degli azionisti e dei risparmiatori sono stati assolti.

truffati da coloro che sono stati ribattezzati «bankster» - metà banchieri e metà *gangster,* con prevalenza dei secondi - che oggi brindano perché questi processi

se questi tribunali sono pronti ad istruire le richieste di giustizia da parte dei cittadini o se ancora non lo sono? Lei viene oggi a rappresentarci una situazione di stato della giustizia con più luci che ombre, e noi, che invece vediamo molte più ombre, abbiamo il dovere di rappresentarlo, perché non è con lo scontro frontale con i magistrati, ma con il dialogo che si cerca di risolvere la questione dei cittadini, di coloro che non hanno diritti, di coloro ai quali i diritti vengono cancellati ogni giorno. È per questa ragione, signor Ministro, che dobbiamo esprimere

quale i diritti possono essere azionabili solo dal 16 agosto 2009, quando la lesione dei diritti risale al 1954? Ritengo che anche quell'azione di classe abbia profili di incostituzionalità, così come

Signor Ministro, sono fortemente deluso della sua Relazione, che per me dovrebbe essere molto importante,

le offrì grande disponibilità, non formale, non a parole. Le offrì il lavoro che era stato realizzato in due anni di Governo Prodi. Il lavoro riguardava l'informatizzazione del sistema integrato giudiziario informatizzato, non la digitalizzazione di questa o quella parte dell'attività giudiziaria.

degli esperti di cui disponeva il Ministero, di tutto il sistema. Lei invece oggi ci ha parlato, con molta - anzi troppa - enfasi, solo delle notifiche, solo delle comunicazioni, tessere importantissime di un sistema che resta non attuato. Non ci ha detto nulla di che cosa è successo in merito al sistema dei registri *web* che lasciammo quasi integralmente realizzato. Non ci ha detto nulla delle banche dati, in parte realizzate e in parte da realizzare, interne al sistema. Che cosa è accaduto delle relazioni e dei collegamenti con le banche dati esterne? Le faccio un piccolo esempio: anagrafe tributaria, banche dati delle polizie, banche dati del sistema bancario. del sistema bancario. Lei sa che il nostro sistema prevedeva tutto questo e che, se attuato, bruceremmo i tempi delle indagini? Un pubblico ministero, collegandosi con quel tipo di banca dati, ottiene risultati di importanti e complicatissime indagini bancarie in pochi ore, non in mesi e talvolta in anni. Questo è tutto nel sistema integrato giudiziario informatizzato che lei avrebbe potuto e dovuto - secondo noi

Signor Ministro, è uno dei punti della nostra collaborazione anche in sede di discussione e di confronto con la sciagurata legge che oggi è stata varata. Se fossero stati accolti i nostri emendamenti, questo provvedimento avrebbe assunto la dignità di legge e avrebbe avuto un senso, un senso, ossia puntare alla riduzione dei processi. Lei ci ha ricordato con molta lealtà che il problema essenziale continua ad essere rappresentato dai tempi del processo. Bene, signor Ministro, con i provvedimenti che ci ha sinteticamente elencato non si abbassano i tempi del processo. Perché nulla è stato fatto in questo settore? Non mi dilungo perché non ho tempo a disposizione, ma potrei citare - per esempio - il sistema già vigente a Napoli che abbiamo introdotto, un sistema meraviglioso che consente il trasferimento delle denunzie della polizia polizia giudiziaria, delle informative già strutturate. Gli addetti ai lavori sanno che cosa ciò significa: quando arriva una informativa voluminosissima già strutturata, viene immediatamente inserita in tutte le procure. Che fine ha fatto il sistema dei fascicoli del pubblico ministero che la procura di Lecce, grazie ai finanziamenti della Regione Puglia, ha attuato da tempo e che andava esteso? Che fine ha fatto l'estensione a tutti i tribunali d'Italia del processo telematico civile relativo al decreto ingiuntivo, operativo a Milano da tre anni? Tutto questo si poteva fare. Perché non sono state realizzate le 26 sale

ma forse ci sarebbe una maggiore condivisione in questo momento fra l'opposizione e la maggioranza: un momento costruttivo che ci è stato impedito dalla rigidità dei tempi): lei ci

Lei ha parlato del momento internazionale. Le ricordo che, prima di lasciare il palazzo in via Arenula, avevamo preparato circa dieci accordi internazionali, bozze pronte per la firma. Quegli accordi con Paesi chiave,

e una serie di attività che agevolerebbero il contrasto al crimine a livello internazionale e alleggerirebbero il peso nelle carceri. Ministro, lei pensa veramente che si possa risolvere questo gravissimo e delicato problema

non ci cita soltanto. Non potrà mai attuare quell'articolo se aumenterà il numero dei poliziotti e lascerà quel numero infimo ed irrilevante di educatori, di assistenti sociali. L'articolo 27 va attuato complessivamente.

del pubblico ministero di svolgere attività dirette a tutelare gli interessi della collettività con la *privacy* e con il diritto-dovere di cronaca dei giornalisti. Questo disegno di legge è pronto: se c'è collaborazione, ci siamo. ci siamo. Sempre per quanto riguarda le intercettazioni, lei sa, perché in quelle circostanze che ho citato glielo ho segnalato ripetutamente, che esiste un sistema che è stato valutato a livello tecnico e scientifico da tre luminari a livello nazionale, che dissero che era un ottimo sistema. Esso consentirebbe

troppe intercettazioni, troppa spesa, è impossibile. Con questo sistema invece la spesa si bloccherebbe e si potrebbe riconoscere quella facoltà-dovere del pubblico

Ministro, la invito a trovare un po' di tempo. Si faccia portare quelle carte. Le analizzi. I suoi collaboratori le devono dare questi risultati perché sono pronti al Ministero. Noi li abbiamo

Signor Ministro, mi permetta di dirle che da quando c'è il Governo Berlusconi si fa un'enorme confusione quando si parla di riforma della giustizia. giustizia. Confusione tra quello che è il piano dell'efficienza dei tempi e della qualità della giustizia e quello del riequilibrio dei poteri volto al ridimensionamento della giurisdizione. L'ambiguità su cui gioca questo Esecutivo è di sovrapporre i due piani senza avere in realtà il coraggio di avanzare serie proposte di riforma. Se si vuole davvero modernizzare la giustizia - e credo che su questo punto siamo tutti d'accordo - occorrono sicuramente una riorganizzazione degli uffici giudiziari, un passaggio effettivo al processo telematico, una semplificazione dei riti, una deflazione delle domande di giustizia, assunzioni, qualificazione del personale e, soprattutto - mi sia consentito, signor Ministro - delle risorse. Cambiare la giustizia si può, riformarla si può, senza però intaccare i principi del nostro ordinamento costituzionale. Invece, per risolvere i problemi della giustizia secondo - mi sia consentito - il pensiero unico di questo Governo, il pensiero Berlusconi, occorre provvedere - ce lo ha ricordato ancora lei oggi in Aula - ad esempio, alla

Desidero poi appuntare il mio intervento sul tema delle sedi disagiate e sui provvedimenti che questa maggioranza ha adottato per risolvere tale problema. Anche se l'ha già

agli emendamenti presentati ieri alla Commissione giustizia della Camera da parte del Governo). Tutto questo perché? Si era pensato di risolvere il problema del riempimento delle sedi disagiate attraverso incentivi economici e di carriera.

dicembre 2009 - assolutamente irragionevole e, anche in questo caso, non inserito in un piano più complessivo, in grado di far fronte veramente alle esigenze di funzionalità ed efficienza degli ufficiali giudiziari

data fra l'altro nella quale non si capisce perché la situazione degli organici degli uffici requirenti nelle sedi disagiate dovrebbe essere diversa da quella disastrosa in cui versa oggi.

anzi, mi correggo, signor Ministro: il Governo Berlusconi si è impegnato in questi due anni a riformare gli strumenti della giustizia che servivano al *Premier*. Anziché scrivere il processo breve, forse avreste potuto fare in termini brevi la riforma della giustizia. *(PD)*. Signor Ministro, durante la sua Relazione ha parlato di una giustizia in crisi: ebbene, credo che si possa andare anche oltre la crisi, visto e considerato che, ad esempio per quanto riguarda le carceri, proprio lei ha parlato di un vero e proprio Piano emergenziale, finalmente presentato in Consiglio dei ministri. Si tratta di una giustizia al collasso, e non lo dicono i radicali, che da trent'anni denunciano tutta una serie di aspetti relativi sia alla violazione dei diritti umani sia alla mancata amministrazione della giustizia, ma la Corte europea dei diritti umani, ieri più volte citata, magari in maniera strumentale, da quello che è stato definito un *mantra*: e lo dice in particolare in merito alla durata dei processi e al modo in cui vengono trattati i detenuti nelle nostre carceri. Sulla prima, avete tentato di rispondere con la legge del cosiddetto processo breve, che nelle prossime settimane vedremo quanto non sarà sufficiente ad affrontare il problema;

che una stragrande maggioranza di coloro che sono in attesa di una sentenza definitiva alla fine del processo viene riconosciuta innocente. Questa è una sistematica violazione dei diritti umani, sanzionata quotidianamente della Corte europea di Strasburgo, che quindi fa diventare l'Italia non più un delinquente abituale, ma un vero e proprio delinquente professionale.

uno dei problemi fondamentali, quello cioè dell'obbligatorietà dell'azione penale che, secondo noi, in questo contesto di giustizia italiana al collasso, e non in crisi, è il problema dei problemi,

adottato durante la scorsa legislatura è stato un pannicello caldo: forse ha ragione. Ci vorrebbe una vera e propria amnistia, che riporti il gioco alla lettera "A" e che dia avvio ad una serie di riforme che ci conducano alla lettera "Z": un'amnistia che

la sua contabilità non tiene conto di tante cose che qui posso soltanto rammentare in modo rapsodico. Analizzando la questione giustizia, si poteva per esempio

Di fronte a questi fatti, che interessano l'intera collettività, il Governo del presidente del Consiglio Berlusconi si è preoccupato ovviamente di prendere provvedimenti che si occupano quasi esclusivamente dei suoi difficili rapporti con la giustizia. Difficili rapporti che hanno ogni tanto degli antidoti isolati. Uno ad esempio, brillantissimo, è la cena inusitata tra il Presidente del Consiglio, lei stesso, signor Ministro, ed altri con due giudici costituzionali,

Invece no. Abbiamo il legittimo impedimento, che serve ad inseguire la prescrizione. Abbiamo il processo breve, che è processo morto, per far fuori il processo Mills, in cui - lo ricordo Mills è stato condannato per corruzione per essere stato corrotto da Berlusconi. Questa è una cosa che non è cancellabile: è lì. Voi volete stabilire una norma che impedisce a Berlusconi di essere riconosciuto come il corruttore di una persona che è già stata condannata per essere stata corrotta da lui.

con una legge di rango costituzionale. Il fatto che sarà una legge di rango costituzionale non eliminerà la violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Tutte le garanzie per gli imputati, tutte le garanzie per l'imputato e nessuna giustizia per le parti lese: questo è uno dei cardini della vostra politica sulla giustizia. Di tutto ci si deve occupare, meno che della giustizia, dell'interesse e dei diritti negati delle parti lese. provvedimento sulle intercettazioni è una perla della vostra pratica sulla giustizia. Esso tronca le indagini, esattamente come il processo breve lo fa diventare un processo morto.

Sono state ingigantite le spese e si dice che le intercettazioni devono essere ridotte. La domanda è semplice: è forse meglio non sapere? meglio non sapere che i mafiosi parlano con i politici? E meglio non sapere che esiste una rete di affarismo ininterrotto tra la politica e la criminalità organizzata? Meglio ignorare? Forse sì, forse è meglio ignorare per la nostra pace mentale, per la nostra pace dei sensi, per la nostra tranquillità. Noi dobbiamo ignorare, meglio non sapere. E questo meglio non sapere si trova anche nei confronti di un aspetto che mi permetto di introdurre qui, anche se so che è leggermente *border line*, perché

aiuti economici solo per i neonati italiani. Ad Alassio (Savona): vietato trasportare merci in buste e sacchi di plastica. E le signore che escono dai supermercati con cosa devono portare via le merci? Ma, si sa, serve per evitare quei mucchi di roba dentro i sacchi di plastica. A Gerenzano (Varese): i cittadini sono invitati a non vendere o affittare casa agli stranieri. Per non sembrare partigiano, parlo anche della Toscana. Nella civilissima Lucca: vietato aprire "kebaberie" e ristoranti etnici in centro. A Prato, che è pieno zeppo di cinesi: vietato aprire "kebaberie", che non credo vendano il cibo prediletto dai cinesi,

che uno degli elementi fondamentali del vostro ragionamento sarebbe che le indagini devono essere affidate agli ufficiali di polizia e che il pubblico ministero deve essere come appartato, separato, messo da una parte;

D'accordo che esiste l'autonomia del politico e che si può pensare che il politico possa essere dotato di un punto di vista superiore, ma arrivare a ritenere di spoliticizzare il Consiglio superiore della magistratura riempiendolo di politici è davvero un capolavoro di retorica. *(Applausi dal Gruppo Signora Presidente, signor Ministro, credo che stasera abbiamo sentito una Relazione sostanzialmente identica a quella dell'anno scorso.

la rivelazione che altrettanto sostanzialmente i problemi elencati l'anno scorso sono rimasti, dal punto di vista della loro soluzione, sul tavolo: non vi è stato un passo in avanti rispetto all'enunciazione delle questioni che abbiamo sentito quindi di fronte allo stesso elenco di problemi dell'anno scorso, senza avere la possibilità di dire (come si sosteneva in un una propaganda politica): fatto. difficile mettere la linea rossa sull'elenco del 2009 rispetto alla Relazione del 2010,

è vero che il recupero crediti da una disputa commerciale nel nostro Paese comporta 1.210 giorni, in Francia 331, in Germania 394;

siamo forse spettatori? Possiamo limitarci a descriverli e a ripeterli annualmente nella loro drammaticità?

sul resto osserviamo una mancanza di risposte, se non una genericità. Mi riferisco ad esempio al tema delle carceri. Un anno fa è stata annunciata la nomina del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria quale commissario straordinario per risolvere l'emergenza carceri. Durante l'anno, in estate e in autunno, si è parlato addirittura di modello Abruzzo,

per le sedi disagiate: dopo un anno il problema è ancora aperto ed i cittadini restano attoniti nel vedere come tale questione, con un conflitto all'interno dello Stato, non ha

«Questo Governo, dunque, procederà alle riforme ordinamentali e processuali che sono necessarie per restituire dignità e credibilità al sistema Giustizia, non certo in ordine sparso ma con un preciso disegno strategico. Per tali ragioni siamo portatori di un approccio globale al tema giustizia

con la concessione di ulteriori termini per la preparazione della difesa, nuove regole sulle prove, istituzione di un tribunale collegiale addizionale per la revisione giudiziaria e la custodia cautelare, nuove regole per l'astensione e la ricusazione dei giudici. di quella proposta di riforma del processo penale, sulla quale ci apprestavamo a confrontarci, si sono perse le tracce. Abbiamo invece visto arrivare improvvisamente tre articoli, e quelli sì hanno riformato il processo penale;

molto difficile parlare di riforme costituzionali o istituzionali condivise. Se non si riesce a ragionare insieme su questioni per certi versi persino neutre, penso che sarà molto più complicato e difficile ragionare su riforme di sistema costituzionale di sistema costituzionale ed istituzionale. Signor Ministro, ho ascoltato con grande attenzione e senza pregiudizi la sua Relazione, ma, vede, questa mattina è stato approvato un provvedimento in quest'Aula che non solo non tutelerà i cittadini italiani, ma determinerà un vero e proprio collasso dell'intero sistema giudiziario. Non c'è dubbio, il problema che colpisce prima di tutto è quello dell'eccessiva lunghezza e farraginosità delle procedure giudiziarie. Si tratta di una questione riconosciuta da tutti gli attori del processo, sia magistrati che avvocati, e da tutti gli osservatori esterni (mondo politico, economisti, sociologi, mondo dell'informazione). Altrettanto certo è che il rimedio a tale situazione patologica non possa non essere strutturale. Occorre ridefinire dalle fondamenta l'organizzazione e la gestione dei sistemi giudiziari italiani, ed occorre farlo in maniera non episodica, ma proficua e stabile. Non ci si può muovere sempre sulle emergenze. Non basta prevedere per legge che un processo non possa durare più di un certo termine ma occorre, altresì, fornire gli strumenti giuridici, economici e pratici perché quei termini (o comunque termini ragionevoli) siano rispettati. In particolare, occorre rivedere completamente le procedure e i riti, tanto quelli civili quanto quelli penali, e occorre farlo, finalmente, in maniera sistematica e non per interventi approssimativi ed episodici. Occorre poi farlo con metodo democratico, non formulando dall'alto ipotesi gradite, ma coinvolgendo nell'analisi critica la magistratura, l'avvocatura, le cancellerie, l'università ed il mondo accademico. Solo in questa maniera, con la predisposizione di progetti di riforma tecnicamente condivisi, si potrà avviare una proficua discussione politica, che porti a riforme concrete discusse e parimenti condivise. A tal proposito, ci chiediamo come la maggioranza intenda affrontare il tema delle riforme costituzionali. Ci auguriamo che lo faccia in maniera condivisa e non in modo autosufficiente. Siamo d'accordo su quanto esposto dal Ministro in merito a procedure più snelle, a termini certi e brevi e al rispetto di un nucleo centrale (minimo e sufficiente) di garanzie per tutte le parti dei processi; efficienza organizzativa, con processi interamente digitalizzati, riduzione del materiale cartaceo, generalizzazione dei sistemi e delle procedure informatiche; riforma urgente del sistema delle notificazioni (enorme falla del sistema giudiziario, che lo stesso Ministro ha ricordato); efficace revisione delle circoscrizioni giudiziarie senza cedimenti campanilistici e con fissazione di limiti minimi, al di sotto dei quali non si potrà mai scendere nella creazione o nel mantenimento di tribunali o procure. Anche l'ordinamento giudiziario merita miglioramenti: certamente il dialogo sul tema della riduzione degli organici delle procure, e più in generale delle cosiddette sedi disagiate, deve essere approfondito, ma non possiamo pensare di usarlo come grimaldello per aprire il sistema di garanzia dell'inamovibilità del magistrato. Ripensare le regole introdotte nel 2006 dalla cosiddetta riforma Mastella, ritornando al sistema di assegnazione a sedi disagiate di procura di magistrati di prima nomina, secondo il meccanismo razionale e ragionevole da noi proposto, è ormai necessario; così come rivedere il quadro dei vantaggi economici e di carriera per i magistrati che prestano servizio in quelle sedi disagiate. Allo stesso tempo, appare utile ripensare in generale alle regole di valutazione dei magistrati, ipotizzando di introdurre sistemi di premialità per la produttività e la laboriosità, insieme al rafforzamento di strumenti di verifica, senza indulgere alla facile demagogia. Queste sono questioni concrete e non secondarie rispetto al tema, sul quale occorre fornire la massima disponibilità alla discussione, della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Nella materia penale è imprescindibile una seria depenalizzazione, perché i tribunali si occupino seriamente delle questioni serie, e non sprechino risorse, tempi ed energie in indagini e processi per reati bagatellari. In questo caso la riforma auspicata è complessiva e di sistema, perché una seria depenalizzazione non può prescindere dalla relativa «copertura amministrativa»: in altre parole, è necessario che il sistema amministrativo complessivo sia tale da fornire comunque una risposta (con controlli e sanzioni amministrative, appunto) alle esigenze sottese alle regole oggetto di depenalizzazione. Il sistema giustizia ha allora bisogno di risorse finanziarie, importanti e costanti, per la modernizzazione delle strutture e delle procedure, per le esigenze di depenalizzazione, per l'aggiornamento e la formazione del personale. Di queste spese si vorrebbe sentire più spesso parlare, e non solo di spese per le intercettazioni. Il Ministro ha riferito sul Fondo unico, ma ha trascurato di precisare che il Fondo unico non compensa quanto è stato tagliato in materia di giustizia in questi anni. Anche la materia del contrasto alle mafie merita un'immutata attenzione: abbiamo appreso con interesse della spinta propositiva del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia alla creazione di un testo unico della normativa antimafia. Occorrono anche in questo caso attenzione e coesione istituzionale, perché l'argomento sia trattato con delicatezza e le scelte legislative siano condivise, nell'ottica di un rafforzamento degli strumenti normativi di contrasto, già rilevanti ed efficienti, come confermato dall'interesse

del sovraffollamento e della vivibilità degli istituti penitenziari sia affrontata seriamente e non con proclami. Si devono, allora, organizzare subito progetti operativi e stanziamenti concreti che possano ovviare in tempi brevi a tale questione. Dichiarare lo stato di emergenza e conseguentemente nominare un commissario straordinario che provveda alla realizzazione di nuove strutture carcerarie è condivisibile, ma non è sufficiente. A nostro avviso sarebbe necessario affrontare il problema, come peraltro abbiamo già detto, ricorrendo alla depenalizzazione dei reati di minore allarme sociale. Infine, nessuna amnesia governativa può riguardare il processo amministrativo, che al momento sfugge alle competenze del Ministro della giustizia. Occorre verificare se si possa parlare di tempi ragionevoli della giustizia senza che ciò riguardi anche i processi amministrativi, in cui i tempi si stanno dilatando anche più delle infinite procedure civili. È forse arrivato il momento di ripensare all'unità, anche amministrativa, della giurisdizione e riformare non solo i codici di procedura amministrativa, ma anche il sistema complessivo di questa giustizia, che appare pronta per una riforma organica.

affrontare il profilo del governo generale del settore della giustizia, la sua cosiddetta gestione strategica, che è reclamata. Un governo del settore che, nella consapevolezza di tutti noi, è difficile e complesso perché porta dietro di sé anche disattenzioni che si sono accumulate nel tempo: pigrizie di carattere legislativo e e dimenticanze di carattere amministrativo che i Governi che abbiamo alle spalle hanno manifestato verso il settore. un aspetto della complessità del sistema che riconosciamo essere fonte di preoccupazione e che in questo tempo iniziale di legislatura noi non abbiamo mancato di segnalare. Dentro un quadro complesso vi sono state e permangono iniziative legislative del Governo e anche del legislatore che che per molti aspetti potremmo definire delle incursioni nel governo del settore che ne accrescono le difficoltà, e soprattutto ne accrescono i tratti di imprevedibilità e quindi di inaffidabilità che, invece, il sistema deve contrastare. Le porto, signor Ministro, per l'attenzione che potrà dedicarvi, due esempi. Il primo riguarda le misure sulla sicurezza. che tali misure sono partite, almeno nelle intenzioni del Governo, da esigenze più specificamente legate all'ordine pubblico,

le condizioni di chi vive in carcere sono disumane e via via gli indicatori della vivibilità nelle carceri collocano il nostro in in una posizione arretrata rispetto ai Paesi occidentali. Cito questo esempio, signor Ministro, per dire che un'azione svolta senza prevederne gli effetti sul sistema giudiziario

me lo consente, signor Ministro, un provvedimento di così vasta portata, capace di determinare effetti così estesi nel settore,

della pena e dell'affidabilità del sistema giustizia nel nostro Paese. Inoltre, in un settore come quello della giustizia, che esige più risorse umane e finanziarie,

non dovremmo consentire più tutti noi che siamo delegati in vario modo ad occuparci del sistema, che avvengano queste forme di incursione. C'è bisogno di una visione strategica e c'è bisogno soprattutto di una gestione responsabile del settore, che noi auspichiamo e che per molti aspetti, purtroppo, non registriamo nella sua Relazione.

tenuto conto di quanto finora ha ascoltato in quest'Aula. Ma voglio rassicurarla: la maggior parte di coloro che siedono nel Senato della Repubblica condivide quanto ha detto, ed è accanto a lei. lei. Ascoltando le sue parole si è percepito nettamente il senso del cambiamento, il passaggio, finalmente anche nel delicato comparto della giustizia, dalla cultura della gestione eterna dei problemi alla cultura del fare. Abbiamo sentito una diagnosi impietosa e, al tempo stesso, scevra da ipocrisie, ma abbiamo sentito anche, per la prima volta, una prescrizione terapeutica che non si tradurrà nell'ennesima grida manzoniana, ma che già ha prodotto risultati e proprio per questo è particolarmente credibile. Ha prodotto risultati in situazioni assolutamente emergenziali, e bene ha fatto, forse con un moto anche di commozione e di orgoglio, a ricordare quanto è stato fatto nella disastrata contrada dell'Aquila per quella città e per tutti gli abruzzesi. Bene ha fatto a ricordare a ricordare che il delicato comparto della giustizia, per vedere finalmente risolta una crisi ormai quasi irreversibile, deve necessariamente tener conto, una volta per tutte, anche e non solo delle risorse finanziarie (che sappiamo essere, peraltro, non troppo dissimili da quelle di altri grandi Paesi europei), ma soprattutto delle risorse umane, e di come congiuntamente risorse umane e finanziarie devono essere impiegate. Quindi, ben venga una cultura manageriale per chi deve dirigere gli uffici, cosicché finalmente questi uffici, che oggi funzionano a macchia di leopardo, con una disomogeneità di funzionamento assolutamente incomprensibile, si allineino. Bene ha fatto il Governo a intervenire in modo concreto per quanto riguarda le sedi disagiate, con incentivi da un lato, ma anche con provvedimenti, se vogliamo, emergenziali e transitori, ma che in qualche modo quel fattore umano dovevano necessariamente responsabilizzare. E debbo darle atto, signor Ministro, a lei come titolare del Dicastero e al Governo che questa maggioranza sostiene, al di là di quello che spesso risuona in questa Aula, forse in modo più scomposto ed offensivo di quanto in realtà il dibattito meriterebbe, di aver saputo trovare un ragionevole *mix* tra iniziativa governativa e parlamentare anche in una serie di provvedimenti in parte già approvati e in parte in corso di approvazione, con un *iter* parlamentare così rapido da non avere precedenti nella storia parlamentare di questo Paese. Abbiamo già riformato il processo civile. Noi, che spesso veniamo accusati di essere una maggioranza oscurantista, in tempi rapidissimi abbiamo approvato quella legge sullo *stalking* le cui cifre applicative ella ci ha già fornito. Noi, che in qualche modo saremmo chissà come collusi con chissà chi, abbiamo promosso la più straordinaria attività legislativa in tema di contrasto alla criminalità organizzata, e i frutti si sono visti in termini concreti. Abbiamo avuto a cuore, noi, gli insensibili, più di ogni altro i problemi della sicurezza dei più deboli in questo Paese perché nel pacchetto sicurezza non solo è stata ribadita la sovranità dello Stato, ma parimenti ci si è preoccupati proprio di tutelare efficacemente e concretamente i più deboli. E se è vero che il valore di un Governo e di una maggioranza si misurano sulle loro iniziative legislative, ebbene, credo che nessuno questo possa negarlo o contestarlo. Il Fondo giustizia, tanto irriso, ha cominciato a produrre i propri risultati concreti e oggi se, grazie anche ad un'intelligente valutazione di carattere emergenziale della situazione carceraria, un Piano carceri finalmente si avvierà, si deve anche a quel Fondo giustizia che oggi ha cominciato a produrre centinaia di milioni di euro per questo comparto. Questo è un altro fatto e, ancora, un altro passaggio della cultura del fare. Mi lasci dire, signor Ministro, in questi pochi minuti che ho a disposizione, che se c'è un passaggio della sua Relazione che più di ogni altro ha convinto chi le parla e ha convinto la maggioranza che siede su questi banchi è stato il richiamo forte alla definitiva attuazione dei principi costituzionali dell'articolo 111 della Costituzione in tema di giusto processo. Il primo passo lo abbiamo fatto in quest'Aula per quanto riguarda la ragionevole durata del giusto processo. Ma bene ella ha fatto a ricordare che il giusto processo si può avere soltanto laddove si abbia un giudice terzo e due parti che si confrontano su un piano di assoluta parità processuale, cosa che in questo Paese ancora è ben lungi dall'essersi realizzata, ed anzi quelle che potevano essere le premesse del codice di rito del 1989 sappiamo bene quanto sono state svilite e sappiamo bene quanta responsabilità abbia anche in questo una parte - forse minoritaria dal punto di vista numerico, ma particolarmente attiva - della stessa magistratura. In questi giorni, in previsione della sua presenza in quest'Aula, durante il dibattito sulla ragionevole durata del processo ci siamo sentiti dire che sarebbe venuto qui a fare il gioco delle tre carte. Dopo aver ascoltato la sua Relazione io le dico: continui a farlo quel gioco, perché nel gioco che lei fa la carta vincente la scopre sempre il popolo italiano.

stiamo parlando della Relazione annuale del Ministro della giustizia: credo che di annualità, di ritualità, nella situazione in cui ci troviamo, davvero non ci sia nulla. Qualche numero lei l'ha fatto e ci tengo a sottolinearlo: 65.774 detenuti ammassati in celle che possono contenerne 43.220, di cui 40.915 italiani e 24.152 stranieri; 800-1.000 nuovi ingressi al mese; 6.261 agenti in meno di quelli previsti in pianta organica; 402 educatori in meno rispetto alla pianta organica; un solo psicologo, per poche ore lavorative a settimana, ogni 187 detenuti;

Solo un detenuto su quattro ha la possibilità di lavorare e solo uno su 10 può partecipare a corsi professionali. Tutti gli altri sono costretti a passare nell'ozio, in celle sovraffollate, dalle 18 alle 22 ore al giorno. Sono 70 i bambini sotto i tre anni carcerati con le loro madri. Il Piano carceri, fosse anche approvato oggi, domani partisse e domani l'altro diventasse realtà, non ci aiuterebbe a risolvere questa situazione. Il totale dei processi pendenti è noto: sono quasi 11 milioni i processi pendenti. Tra la data del delitto e quella della sentenza la durata media è di 35 mesi per il primo grado del processo e

Credo che solo un provvedimento dovrebbe avere l'onore del dibattito di queste Aule parlamentari e solo un impegno del Governo e del Parlamento potrebbe davvero farci uscire da questa situazione di ingiustizia, di violazione dello Stato di diritto: si chiama amnistia. Signora Presidente, signor Ministro della giustizia, colleghe e colleghi, dobbiamo cominciare a credere nelle fortunate congiunzioni astrali perché, evidentemente, non può essere casuale che ella, Ministro, venga oggi in questa stessa Aula del Senato in cui, in sua assenza, la maggioranza a sostegno del Governo cui lei appartiene ha approvato una delle più brutte leggi della storia repubblicana: il cosiddetto ammazza-processi, un provvedimento che, stando alla concorde lettura delle fonti di informazione e alle dichiarazioni di tutti gli interessati, è stato fortemente sostenuto dal Governo, da lei stesso e dagli avvocati del Presidente del Consiglio e che, per i suoi molteplici profili di irragionevolezza e palese incostituzionalità, si configura tale da infliggere al sistema giustizia nel suo insieme e a quello giurisdizionale in particolare un colpo catastrofico se venisse approvato anche alla Camera. Non lo dice l'opposizione, non lo dice quel pericoloso soggetto eversore che è l'Italia dei Valori, ma lo gridano a voce alta il Consiglio superiore della magistratura, il Consiglio nazionale forense, le Camere penali, l'Associazione nazionale magistrati. Lo dicono sommessamente molti parlamentari della stessa maggioranza. Eppure, Ministro, l'efficienza del sistema giudiziario e l'accelerazione dei processi (non la loro morte), la rapidità dell'accertamento dei reati e la conseguente certezza delle sentenze e dell'espiazione della pena dovrebbero costituire la principale occupazione e preoccupazione del Ministro della giustizia e del Governo nella sua collegialità. Si assiste invece a scelte che, dal punto di vista delle politiche finanziare, delle dotazioni infrastrutturali, del mancato potenziamento delle risorse umane e dello squilibrato quadro normativo, non vanno in quella direzione. Per questo, Ministro, ci vuole un bel coraggio e - se mi permette - una bella faccia tosta ad aver scelto proprio la giornata odierna e proprio il Senato per propinarci il regno del bengodi: una giustizia pronta e tempestiva, nuova e moderna che, con un colpo di bacchetta magica, nel corso del 2010 ella riuscirà a rimettere in sesto. Ce lo auguriamo per gli italiani! lo vogliamo augurare per gli italiani, perché la riforma della giustizia sta a cuore a lei, a noi e a ogni cittadino che vuole vedere riconosciuto un diritto, ma che vuole anche poter aver le sentenze Invece, con un colpo di cipria lì, un *lifting* là e una maschera carnascialesca qua si cerca, se non di nascondere, di dipingere a tinte rosee una situazione drammatica che il Governo a cui lei appartiene, anche in questo scorcio di legislatura, ha contribuito sistematicamente ad aggravare. Ministro, una delle questioni cruciali per il nostro Paese è rappresentata dalla risposta che il sistema giustizia è in grado di offrire al fenomeno della corruzione che, oltre a determinare sacche di diffusa illegalità, costituisce una zavorra per lo sviluppo e il progresso economico e sociale, oltre che una scorciatoia verso fenomeni di vera e propria immoralità e di disincentivazione degli investimenti stranieri. Su questo concordiamo con lei, ma il dover pagare mazzette - altro che ulteriori balle - è il vero motivo del disinteresse dei capitali stranieri in Italia e nel Mezzogiorno in particolare. È evidente che una risposta a tale problema non investe solo il piano giudiziario. Occorre, infatti, ricordare che il Consiglio d'Europa ha più volte sottolineato criticamente come proprio la prescrizione dei reati incida pesantemente sui processi per corruzione, su quelli di criminalità, invocando riforme che consentano di addivenire alle sentenze di merito, quelle sentenze a cui non si arriva mai. Le riforme che ci vengono invece proposte dal centrodestra con il suo autorevole avallo, sovrapponendo la prescrizione dei processi a quella sostanziale del reato, rendono più difficile, a giudizio dell'avvocatura associata e della magistratura, l'impegno dell'Italia nella lotta alla criminalità, e alla corruzione in particolare, reato per il quale la prescrizione breve ha purtroppo dispiegato i suoi effetti. di Stati contro la corruzione ha inviato all'Italia ben 22 raccomandazioni per evitare la morte dei processi: proprio quello che questa mattina voi invece avete votato. Noi vogliamo pronunce, pronunce vere. Ecco perché abbiamo presentato fin dal maggio del 2008, pochi giorni dopo l'insediamento di questa legislatura, 25 disegni di legge che vanno verso una riforma complessiva della giustizia. Altro che dire sempre no! Abbiamo cercato di riorganizzare, di offrire soluzioni, ma nelle Commissioni questi disegni di legge sono nel cassetto. Perché? Perché bisogna discutere del lodo Alfano, lodo che sciaguratamente porta il suo nome e che sappiamo che fine ha fatto.

sempre ed esclusivamente i problemi del suo Presidente del Consiglio, il Presidente del partito dell'amore *(Applausi dal Gruppo IdV)* che oggi ha dichiarato che non va a farsi giudicare perché i suoi avvocati hanno detto che andrebbe davanti al plotone d'esecuzione.

di chi scappa davanti alla giustizia! Siamo disponibili, sappiamo che ci sono dei problemi e li vogliamo risolvere: l'informatizzazione, la riduzione dei formalismi che ritardano e spesso fanno caducare i procedimenti,

senatore Li Gotti nella sua dichiarazione di voto, ricorderemo all'Aula su quali contenuti vogliamo le riforme.

su tutte le richieste e i diritti dei cittadini italiani. Invece abbiamo la speranza che, come San Paolo sulla via di Damasco, anche i peccatori più incalliti cambino orientamento cambino orientamento e si seggano a ragionare su quello che serve al Paese e non su quello che serve alla vostra maggioranza e al Presidente del Consiglio.

Questo per due ragioni: la prima è che è bravo, la seconda è che è anche fortunato perché ha alle spalle la maggioranza più coesa e più forte che ci sia mai stata in un Parlamento della Repubblica. Questo semplicemente perché - non me ne voglia l'ex ministro Castelli, che ha fatto tutto quello che poteva in un periodo molto difficile - in questo momento la semplificazione del quadro politico e il fatto che la maggioranza sia composta da due soli partiti,

È chiaro che questo dà molto fastidio. Signor Ministro, lei è inoltre fortunato per un'altra cosa: perché viene a portare la sua Relazione sullo stato della giustizia poche ore dopo l'approvazione in quest'Aula di un importantissimo provvedimento in materia. Abbiamo approvato finalmente la riforma sui processi brevi.

A questo punto, il provvedimento va bene se non produce effetti nei confronti di una persona, ma non va più bene se produce qualche effetto (e sappiamo chi è la persona al centro di ogni disputa politica). I nostri maestri dottrinari, signor Ministro, dai quali abbiamo praticamente attinto tutti nella nostra formazione, ci hanno sempre ripetuto che una giustizia non tempestiva non può nemmeno dirsi giustizia.

non arriveremo a commentare tutto quanto ha elencato il Ministro tra le cose fatte e gli impegni che il Governo e il suo Ministero hanno

dai genitori o leggendo quel poco che hanno potuto leggere - cosa stava accadendo nelle Aule del Parlamento. Il Ministro ha annunciato un intervento estremamente razionale: un piano di edilizia penitenziaria, con 47 nuovi padiglioni e

ha messo in luce che questo è forse il Governo più efficiente che il Paese abbia mai avuto. Esso ha affrontato un'emergenza in modo impeccabile, tempestivo e risolutivo: non si era mai vista una cosa del genere.

Concludo con l'affermazione che ha fatto il nostro collega capogruppo Bricolo. Abbiamo un periodo favorevole: per tre anni non avremo l'incubo di elezioni; e noi sappiamo come le elezioni condizionino il dibattito in quest'Aula. Non ci saranno esasperazioni di toni e, probabilmente, le contrapposizioni strumentali saranno ridotte al minimo, mentre oggi invece esplodono.

ricca di aggettivazioni enfatiche in molti punti. Ho constatato, in particolare, l'uso ripetuto della parola "straordinario" nella sua accezione positiva, riferita alla sua personale attività di governo, signor Ministro, e all'attività della compagine di cui lei fa parte. I toni declamatori e trionfalistici della sua Relazione appartengono allo stile della comunicazione politica, sul quale naturalmente possiamo avere le nostre opinioni, ma che non è l'oggetto specifico della riflessione che dobbiamo La questione, purtroppo, è che certamente ci troviamo in una situazione straordinaria e di fronte ad un'azione straordinaria della compagine governativa di cui lei fa parte, della maggioranza cui lei fa riferimento e del suo stesso Dicastero. La direzione, però, e il senso della straordinarietà non sono - temo - nel senso e nella prospettiva da lei indicate. C'è un lancio dell'ANSA di oggi pomeriggio, in cui non le minoranze di magistrati politicizzati (cui fate riferimento senza mai specificare a chi effettivamente intendiate alludere), ma il Comitato intermagistrature (cioè la magistratura ordinaria, la magistratura contabile e la magistratura amministrativa) che con il disegno di legge sul processo breve verranno posti nel nulla centinaia di migliaia di processi, con un costo sociale ed un danno erariale altissimi. È la questione del denaro, di cui lei bene ha fatto a parlare riferendosi alle intercettazioni, signor Ministro, Sono destinati all'immediata estinzione - lo sapevamo tutti, ma giova ripeterlo - i reati contestati nei processi per i *crac* Cirio e Parmalat, per le scalate alle banche Antonveneta e BNL, per la corruzione nella vicenda ENI Power, per le morti bianche alla ThyssenKrupp, per le morti di amianto.

i parenti delle vittime della ThyssenKrupp, i parenti delle vittime dell'amianto, le persone gettate sul lastrico dai *crac* Cirio e Parmalat. Questo sarebbe il minimo necessario per sostenere con dignità questo punto di vista. le altre cose lei ha fatto riferimento, nel suo intervento, alla materia delle intercettazioni, rivendicando al suo Dicastero una riduzione delle spese per le intercettazioni a seguito di una bonifica contabile, della quale naturalmente ci compiacciamo. Io presumo che lei sappia come funziona il meccanismo delle tariffe in base al quale noi tutti paghiamo le intercettazioni: funziona essendo collegato alle tariffe che attualmente sono ordinarie da parte dei gestori di telefonia che sono concessionari di servizio pubblico. Sono certo che lei lo sa, ma lo ricordo a tutti quanti: negli altri Paesi, al momento del rilascio della concessione, vengono definite tariffe speciali per le intercettazioni (quindi per lo Stato), operazione che di per sé sola Così come abbattimenti di spese ben più significativi di quelli da lei rivendicati avrebbe consentito o consentirebbe, se lo si volesse, l'adozione del meccanismo di cui ci ha parlato il senatore Maritati. So di avere poco tempo, quindi davvero desidero attirare l'attenzione sua e sua e della maggioranza, rappresentata sinteticamente (così come la minoranza) in quest'Aula in questo momento. Abbiamo un disegno di legge sulle intercettazioni, che avete approvato alla Camera, cui si fa riferimento per alludere a un nuovo sistema di garanzie, oltre che a un meccanismo di riduzione della spesa. Vorrei raccontare in termini molto sintetici una delle possibili conseguenze dell'approvazione, ove dovesse verificarsi anche qui, di quel disegno di legge in quei termini, un esempio tra i tanti per dare l'idea della schizofrenia normativa cui stiamo assistendo. Mi riferisco ad un'indagine in materia di stupefacenti, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti:

a un reato di sequestro di persona, stupro e omicidio di un bambino che non ha nessun collegamento probatorio e nessuna forma di connessione con l'attività di traffico di stupefacenti per cui si indaga. In base a elementari criteri di ragionevolezza, nell'attuale sistema quella intercettazione, in cui viene confessato un reato di eccezionale gravità, sarebbe utilizzabile; invece nel sistema delineato

contiene anche cose esatte e che possiamo condividere (poche), ma nel momento in cui registravo alcuni degli aspetti su cui possiamo essere d'accordo, che per lo più sono il recupero di prodotti legislativi della precedente legislatura, mi viene in mente una famosa e bellissima metafora. Sa, signor Ministro, qual è l'orologio che segna l'ora più esatta di tutti, l'orologio di maggior precisione e il più funzionante

Signora Presidente, colleghi senatori, onorevole Ministro, io desidero invece complimentarmi con lei per una Relazione che illustra il lavoro svolto e prepara il futuro. il primo dei quali concerne la parte del lavoro svolto con l'intelligenza di aver razionalmente capito che per aggredire la criminalità organizzata in questo Paese bisognava finalmente prendere atto, anche dal punto di vista legislativo,

chiudere il buco nero nella storia della Repubblica rappresentato da quelle stragi sarà ben spesa da tutti i magistrati che lo fanno, a condizione che lo facciano per darci verità e giustizia),

mafia aveva bisogno di una legislazione nuova, che qui è stata posta in essere, sotto il suo impulso, con la collaborazione di un Parlamento che in questo caso, rompendo le pregiudiziali, è riuscito a dare un contributo complessivamente positivo nel settore dei sequestri e delle confische dei patrimoni, con il carcere duro inasprito al punto da provocare reazioni terribili, con il potere di accesso dei prefetti nei cantieri, con la nuova norma sullo scioglimento dei Comuni che prevede anche la possibilità di perseguire i dirigenti e non soltanto il ceto politico; con l'inizio di una nuova legislazione sul riciclaggio, che è la nuova fronte frontiera di questa norma. Onorevoli senatori, gli esperti ci insegnano oggi che una massa di denaro può essere lavata (come si dice in gergo) 80 volte in 24 ore senza lasciare traccia di sé e questa è la nuova frontiera della lotta per la legalità in questa e nelle altre democrazie occidentali.

che riguardano la nostra Costituzione in materia di giustizia. Voglio dirle, Ministro, che il Parlamento è qui per cercare di aiutare tale percorso aprendo un dialogo con tutti i soggetti istituzionalmente interessati. interessati. Stiamo infatti per avviare un ciclo di audizioni in cui potremo confrontarci con le alte cariche della magistratura, con le associazioni dei magistrati,

senza che quello che chiamate consenso quando prendete i voti, diventi deriva plebiscitaria quando i voti li prende Berlusconi, il quale non sta al suo posto se non perché da quindici anni è il cittadino più votato da milioni di italiani, e si assume responsabilità di governo che gli vengono assegnate dal popolo con libere e segrete elezioni. Chiamatelo come volete, ma io non conosco altro modo di vivere la democrazia se non rivolgendosi al popolo; né mi convince la teoria degli intellettuali che parlano di «popolo bue» quando non vince la sinistra, perché non mi è mai piaciuta questa interpretazione dei fatti. dei fatti. Possiamo aprire un dialogo a una condizione: che ci siano soggetti che vogliano interloquire fra di loro per cambiare il sistema e fare le riforme istituzionali, sapendo che tutti, non soltanto i magistrati ma anche la politica, debbono essere indipendenti nella possibilità di svolgere il loro compito, per ristabilire un rapporto tra le istituzioni che rappresenta l'equilibrio politico-istituzionale su cui vive la nostra democrazia. Dal momento che sulla suddetta strada lei, Ministro, ha avviato non solo un confronto, ma un'apertura per ragionare sulla giustizia del futuro, la ringraziamo per essere venuto in questa Assemblea, come lo scorso anno, con un bagaglio di cose fatte e con il progetto delle cose da fare. Siamo pronti a darle la piena disponibilità per accompagnarla nel difficile ma esaltante compito di riformare la giustizia italiana.

prevalentemente costruttivo, una volontà di realizzare quelle riforme della giustizia che sono alla base della speranza di cambiamento del sistema giustizia in Italia. Quasi tutti gli interventi sono stati tendenti comunque a porre in essere proposte e suggerimenti. Ho letto con attenzione tutte le proposte di risoluzione e sono consapevole del fatto che talune, anche per esigenze di tempo,

presentata dal senatore Pistorio e altri, adottando un criterio di prevalenza: al terzo punto di tale proposta, infatti, non condivido l'idea di assumere un impegno per la revisione delle circoscrizioni, perché non ho intenzione di procedere

dal punto di vista della solennità dell'impegno parlamentare non mi sento, con grande serietà, di assumere questo impegno, anche perché ritengo che lo sforzo che stiamo facendo potrebbe sì avere un compimento in una razionalizzazione

giustizia esercitata con efficienza in uffici giudiziari minori e ho visto giustizia esercitata con minore efficienza in uffici giudiziari maggiori: è una questione che va ponderata bene. Secondo il CSM sarebbero ben 88 gli uffici da chiudere; io non condivido questa posizione, ma ci sarà tempo e modo per discuterne. Tornando alla proposta di risoluzione del senatore Pistorio ed altri, ribadisco il mio parere favorevole secondo un criterio di prevalenza, non condividendo,

del presidente Gasparri, del presidente Bricolo e di altri. Vorrei argomentare queste mie considerazioni sulle proposte di risoluzione, sviluppando una breve riflessione di sintesi sul dibattito svoltosi. Ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi devo dire, specificatamente ai colleghi dell'opposizione, taluni dei quali assenti in questo momento, che, avendo anch'io fatto in varie stagioni parlamentari della mia vita, sia nell'Assemblea regionale sia alla Camera dei deputati, il deputato di opposizione, ritengo di poter dire, con consapevolezza, che l'opposizione è tanto più credibile nell'affermare le cose che il Governo non ha fatto quando ha il coraggio e l'onestà di riconoscere le cose che il Governo ha fatto. Mi riferisco a talune nostre iniziative che sono abbastanza certificate agli atti, ad esempio alla diffusione nel nostro Paese, in questi dodici mesi, dei modelli di autoanalisi e di miglioramento (le cosiddette *best practices*) negli uffici giudiziari. Mi riferisco altresì all'intervento del senatore Carofiglio in materia di intercettazioni, che spiegava come tutte le intercettazioni si possano fare gratis, ma che ha omesso di ricordare a quest'Aula, che pure ha approvato la finanziaria poche settimane fa, che questo Governo, con forza e con coraggio, ha reso per legge obbligatoriamente gratuita l'attribuzione dei tabulati, con un risparmio di spesa di 18 milioni di euro. avrebbe potuto, a sua volta, ricordare gratis l'approvazione di tale misura: sarebbe stato un riconoscimento nei confronti di un'azione di buona gestione della cosa pubblica, approvata peraltro da quest'Aula poche settimane fa e che non si è avuto, non la generosità, ma quanto meno l'onestà, di ricordare. Ciò avrebbe reso più credibile l'intero discorso. In materia di intervento sulle sedi sgradite ai magistrati avrei gradito, a maggior ragione in connessione con un dibattito che alla Camera ha portato ad un voto all'unanimità, il riconoscimento che, a fronte della preesistenza di un problema, c'è stato un decreto

senza incorrere in reprimende; credo che questo migliorerebbe il dibattito e renderebbe anche più concretamente fattiva la collaborazione, che parte dal riconoscimento di talune cose fatte. Oppure, in ambito amministrativo, si può ricordare che dopo dieci anni è stato firmato un contratto collettivo nazionale integrativo del personale dirigenziale del Ministero della giustizia, giustizia, o che si è celebrato un G8 Giustizia, che ha concluso affermando che la piattaforma italiana di contrasto alle mafie è quella accolta come base dalle grandi potenze del mondo come linea di contrasto alle mafie. O riconoscere che nella riforma del processo civile vi erano istituti mutuati da taluni ordinamenti, a cominciare da quello francese dell'*astreinte*, che consentono al giudice di dire: «Caro cittadino, questa è la tua condanna e, se sei inadempiente, questa è la tua penale, che decorre giorno per giorno». Questa legge ha dato maggiori certezze e i nostri giudici l'hanno già applicata.

arrestate 942 persone; o ancora che le misure di prevenzione antimafia hanno prodotto effetti, perché già applicate. E qual è il miglior canone di valutazione di una legge approvata dal Parlamento se non quello del suo immediato utilizzo da parte dei magistrati? Quando una legge non c'è e poi viene approvata e i magistrati la utilizzano subito vuol dire che se ne sentiva la mancanza. Gli esempi che ho fatto sono di leggi approvate in questi ultimi 12 mesi di cui evidentemente si sentiva la mancanza e che i magistrati italiani hanno già utilizzato. Come non ricordare, poi, che alcuni mesi fa, quando lanciai a livello europeo il tema di un'Europa che non può chiudere gli occhi rispetto al sovraffollamento nelle carceri dei Paesi dell'Unione derivante dalla presenza di detenuti stranieri, mi fu rimproverato, con tono solenne, che l'Europa non aveva competenze in materia? Io, senza solennità alcuna, obiettai che non stavamo parlando in materia europea di tavole evangeliche,

dell'opposizione italiana), che insieme ha convenuto la presentazione di una risoluzione al Parlamento europeo; quella risoluzione, dovuta ad una battaglia puramente politica del Governo italiano, sostenuta dall'intera delegazione senza badare ai partiti,

Questi sono risultati ottenuti grazie ad un'azione amministrativa di governo, ad un'azione legislativa in Parlamento e ad un'azione politica in Europa. Questi sono risultati!

È stato necessario che arrivassimo noi per far sì che ci fosse un Governo delle buone leggi, della buona amministrazione e delle buone prassi.

una diagnosi abbastanza condivisa sui mali della giustizia e una terapia sufficientemente non condivisa in materia di soluzione dei problemi: se il parere sulla terapia fosse unanime, voteremmo tutti allo stesso modo e non ci sarebbero distinzioni tra di noi.

abbiamo scelto questa seconda strada - lo dico alla collega senatrice Poretti - accogliendo proposte provenienti dalla Camera, dal PD, dai radicali in primo luogo e anche dalle nostre forze di maggioranza;

nei confronti del sistema carcerario, ma dell'intero sistema del processo penale italiano. Contemporaneamente a questo, abbiamo deciso che se vogliamo risolvere il problema senza mandare a casa

Allora, abbiamo deciso di affrontare di petto la questione e di offrire, per la prima volta, al nostro Paese la possibilità di risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri senza ricorrere all'amnistia e all'indulto, ma ampliando il numero dei posti, e di farlo con procedure straordinarie, anche perché è impossibile immaginare la funzione rieducativa della pena e la dignità della persona in una cella sovraffollata. Quindi, l'edilizia carceraria è parte del percorso di restituzione piena della dignità ai nostri detenuti. Ed ancora, sulla materia dell'arretrato civile i numeri che ho esposto dicono con evidente chiarezza una grande verità: noi possiamo fare in modo che vi sia maggiore efficienza nel nostro sistema

e l'*output,* cioè quanto il sistema del processo civile ne riesce a tirar fuori, si riduca allo zero per cento; quindi 5 milioni ne potrebbero entrare e 5 milioni ne potrebbero uscire. premesso, abbiamo sempre 5 milioni di arretrato alle spalle: il vero zaino di piombo che impedirà al sistema della giustizia civile di correre anche in presenza delle migliori riforme, della più efficace informatizzazione e della più efficace digitalizzazione, quanto un sistema che ha prodotto un accumulo negli ultimi 30 anni di 5 milioni di processi non li può smaltire, se non con modalità straordinarie. Ed è a modalità straordinarie che pensa il Governo, secondo un binario parallelo, che da un lato mette in campo riforma del processo civile e l'efficienza del sistema attraverso una migliore organizzazione degli uffici ed una più efficace informatizzazione e digitalizzazione. Per altro verso, se noi non accompagniamo tutto questo con con un piano straordinario di smaltimento dell'arretrato civile, qualsiasi sforzo per la prospettiva sarà negletto dalla presenza dei 5 milioni di cause pendenti. Questa è la nostra diagnosi sul sistema del processo civile. Ed ancora, sulla scia dei meccanismi di organizzazione. Non esiste nessuna organizzazione complessa - e tale è il sistema giustizia - che possa considerare una variabile marginale, laterale e trascurabile la variabile umana. Noi abbiamo la necessità di porre al vertice degli uffici giudiziari non tanto e non solo raffinati giuristi, quanto abili, bravi, efficaci organizzatori di uomini e mezzi, perché non è possibile che a parità di leggi vi siano tribunali che vanno bene ed altri che vanno male. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).* E non è il destino che condanna taluni tribunali ad andare male rispetto ad altri che vanno bene: è la capacità degli uomini di governare processi complessi ed organizzazioni complesse come quelle di un ufficio giudiziario. Questa è la variabile sulla quale si intende lavorare e, senza voler essere sacrileghi nei confronti dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, ci vuole un di più di meritocrazia, un di più di efficienza, un di più di gestione manageriale degli uffici, che in questi anni non abbiamo scorto se non in talune rispettabilissime eccezioni. Infine, e mi avvio a concludere, questo 2010 secondo noi è l'anno decisivo per la riforma costituzionale in materia di giustizia. La riforma costituzionale in materia di giustizia occupa il dibattito di addetti ai lavori e dell'opinione pubblica da oltre un ventennio, ben prima dello scoppio di Tangentopoli.

e questa nostra maggioranza, avendo innanzi a sé la prospettiva di una legislatura completa, non si farà sfuggire l'occasione di porre mano alla riforma costituzionale in materia di giustizia secondo le linee direttrici che ho trattato poc'anzi. che la riforma della giustizia sia una grande sfida e allo stesso tempo un grande crinale che separerà la voglia di cambiamento dallo *status quo*. Noi in quest'Aula siamo qui a ribadire che ci schieriamo con forza dalla parte del cambiamento, nella consapevolezza che se c'è un modo per non migliorare la giustizia è quello di lasciare tutto com'è, quello di non porre mano alla Costituzione, all'organizzazione e a buone ed efficaci leggi.

Signora Presidente, signor Ministro, siamo convinti che sul tema della giustizia la regola debba essere il dialogo e il confronto. Il sistema giudiziario italiano richiede cambiamenti sostanziali. L'impopolarità di cui esso gode presso l'opinione pubblica sta a dimostrare l'urgenza di seri interventi riformatori. La soddisfazione dei diritti dei cittadini è infatti elemento di misurazione del grado di civiltà di una società. Fra gli interventi più urgenti vi sono, nel settore civile, una razionalizzazione che incida sulla pluralità dei riti, l'adozione del giudice monocratico per il primo grado, la creazione di un unico rito di cognizione, l'assunzione della prova in contraddittorio davanti a un giudice terzo, l'ampliamento della sfera della risoluzione extragiudiziale delle controversie, mutuando, ad esempio, il sistema previsto per gli arbitrati nel giudizio del lavoro, la revisione del sistema impugnativo. Nel settore penale, sono prioritari interventi come la riforma degli istituti della contumacia e delle notifiche, nonché una importante opera di depenalizzazione e di riscrittura completa delle regole del rito. È inoltre necessario che provvedimenti fortemente intrusivi della libertà personale siano tendenzialmente oggetto di una valutazione da parte di un giudice collegiale. Occorre un confronto sereno e scevro da contrapposizioni politiche sul delicato tema delle intercettazioni telefoniche ed ambientali: appare opportuno che le intercettazioni siano disposte anche attraverso la valutazione di un organo collegiale e le spese siano limitate attraverso la predisposizione di centrali uniche di spesa per noleggio di apparecchiature e convenzioni con i gestori di telefonia. È necessario comunque introdurre elementi che, nel rispetto della libertà di informazione, contrastino, anche con l'applicazione di sanzioni pecuniarie interdittive, la pubblicazione arbitraria di documenti giudiziari coperti da segreto. Le misure messe in campo nella lotta alla mafia dal Dicastero sono senz'altro positive, ma sarebbe necessario ad esempio, nell'introduzione di nuove figure di reato, fare valutazioni di coerenza con l'intero sistema. Per questo è apprezzabile la proposta di stendere un testo unico in materia, al cui esame critico e propositivo non ci sottrarremo. È evidente che noi siamo aperti al confronto anche sul tema delle riforme costituzionali. Dal nostro punto di vista, infatti, il tema della riforma costituzionale della giustizia deve essere affrontato, non a pezzi, bensì pensando e costruendo un sistema che stia in equilibrio e che crei un nuovo equilibrio che Signora Presidente, per queste ragioni voteremo contro la proposta di risoluzione presentata dal collega Gasparri e dagli altri colleghi di maggioranza. Voteremo invece ovviamente a favore della nostra e delle altre proposte di risoluzione presentate dal Partito Democratico, dall'Italia dei Valori e dal collega Pistorio. Signor Presidente, signor Ministro, la sua Relazione è francamente deludente. È modesta ed è imbarazzata

che è motivo di profonda irritazione, visto che da un anno chiediamo che venga a riferire in Commissione e invece si sottrae al confronto),

che sono affluiti nel Fondo unico giustizia un miliardo e 590 milioni di euro, ossia

E poi, signor Ministro, non ci venga a dire che si tratta di soldi che vanno alla giustizia, per la semplice ragione

il Governo ha fatto un'altra cosa e lei dovrebbe saperlo, Ministro: ha stabilito che i soldi che vanno a finire nel Fondo unico giustizia verranno suddivisi fino ad una quota del 30 per cento fra tre soggetti: un terzo all'Interno, un terzo alla Giustizia e un terzo all'erario. Quindi, del miliardo e 590 milioni di euro, alla giustizia andranno 159 milioni,

Ha parlato poi delle carceri. «Sul piano dei rimedi, occorre procedere con il piano di edilizia carceraria per la realizzazione di nuove carceri ma anche - e più rapidamente - con l'ampliamento degli istituti penitenziari già esistenti (poiché si registra un tempo medio di tre anni, dall'assegnazione dei fondi alla realizzazione e inaugurazione della struttura), oltre che con l'impiego di ulteriori unità di personale».

É passato un anno e mezzo e ci ha ripetuto le medesime frasi. Che fine hanno fatto i circuiti carcerari virtuosi che lei aveva annunciato, signor Ministro? Che fine hanno fatto? Signora Presidente, non intendo concludere il mio intervento se il Ministro viene distratto. Signor Ministro, che fine ha fatto la politica dei braccialetti elettronici da lei annunciata? È vero o non è vero che il Ministero della giustizia paga ogni anno a Telecom 11 milioni di euro per un unico braccialetto elettronico in funzione ed è impegnato a pagare questa somma sino al 2011? Mi dica, è vero o non è vero? dica se è vero o non è vero. Su queste cose doveva rispondere, Avendo noi formulato delle rituali interrogazioni e non avendo avuto risposte dopo mesi, torniamo sull'argomento. Il dato è stato denunziato dall'Organizzazione della polizia penitenziaria. Lei ha annunciato l'assunzione di 2.000 agenti di polizia penitenziaria. È vero o non è vero che le attuali scoperture ammontano a 5.000 agenti? Il personale amministrativo: è vero o non è vero...

faccia zittire i somari!

anno: visto che nella sua Relazione non parla di questo problema, in che modo si ritiene di risolvere tale problema? Ugualmente merita la nostra totale recriminazione il fatto

invocata per contrastare la mafia. È passato un anno e, nonostante le nostre insistenze in Commissione, non riusciamo a farla andare avanti. Ci sarà poi un motivo per cui il personale amministrativo ha proclamato lo stato di agitazione; la magistratura ha proclamato lo stato di agitazione; l'avvocatura ha proclamato lo sciopero per i giorni 27, 28 e 29 gennaio per protestare contro la politica della giustizia di questo Governo. Signor Ministro, si è chiesto perché queste tre componenti (personale amministrativo, magistratura e avvocatura)

ha abdicato al suo ruolo nel momento in cui, pur essendo Ministro della giustizia, ha ritenuto di dover esprimere giudizi che spettano alla magistratura sul collaboratore di giustizia Spatuzza: non doveva farlo,

Spetta alla magistratura esprimere giudizi, mentre lei, con la buona compagnia del sottosegretario Mantovano, si è divertito Per tutte queste ragioni, esprimiamo un giudizio contrario alla sua Relazione, un giudizio duro come dura è stata la Corte costituzionale verso quella legge che porta il suo nome e sulla quale lei ha glissato, non menzionandola nella sua Relazione. La sua prima legge è stata sonoramente

la giustizia ha il merito - o forse il demerito - di riportare anche in quest'Aula toni un po' più aggressivi.

Signor Ministro, lei giunge in quest'Aula poche ore dopo l'approvazione di un provvedimento importante, che è quello sul processo breve; un provvedimento ispirato alla volontà di rispondere al problema, reale e oggettivo, della durata interminabile dei nostri procedimenti giudiziari, sia civili che penali, con la volontà quindi di riconoscere al cittadino una giustizia certa e non denegata. Ebbene, perché questa scelta, che oggi quest'Aula ha condiviso approvando il provvedimento, sia pienamente credibile, perché sia credibile la scelta del Governo di compiere tutte le iniziative utili a velocizzare e a rendere efficace il sistema giustizia, e per non lasciar intravedere altre finalità in queste scelte, occorre che l'azione dell'Esecutivo si dispieghi

una iniziativa del Governo, e del suo Dicastero in particolare, sulla formazione dei magistrati. Vi era nella legge Mastella una scelta in questo senso, ma essa è rimasta inevasa. Io credo che la professionalità dei magistrati e la loro capacità siano le migliori garanzie di autonomia e di indipendenza. Quindi una scuola di formazione per la magistratura è per noi un punto irrinunziabile. dalla scelta di caricare sui vertici degli uffici giudiziari il compito organizzativo *lato* *sensu*. Appare infatti inappropriato, per la formazione giuridica che deve presiedere ed assistere costoro, caricare i vertici di responsabilità gestionali che muterebbero in modo troppo profondo la loro connotazione. Soprattutto, quando questo diventa elemento valutativo predominante nella scelta degli incarichi dirigenziali, rischiamo di non avere più

che superi la vecchia e antiquata dimensione del cancelliere e gli faccia carico delle responsabilità logistico-organizzative in termini gestionali, possa essere - quella sì - una separazione delle attività e delle funzioni corrispondente agli interessi del sistema. È necessario che i magistrati vengano giudicati sulla

delle sedi disagiate è legato, oltre che ad alcuni meccanismi legislativi che abbiamo condiviso, ma che portano ad alcuni eccessi di rigidità nel regime delle incompatibilità (che potrebbe essere oggetto secondo noi di qualche intervento modificativo, riducendo l'incompatibilità regionale a livello distrettuale),

razionale in termini di sedi giudiziarie improduttive o troppo decentrate. Un altro aspetto che condivido della sua impostazione è la decisione di abbassare il flusso di accesso al sistema giurisdizionale sia per la sede civile che per quella penale. Da una parte dovrà essere sviluppata l'area arbitrale e l'area della conciliazione, anche utilizzando sedi innovative di conciliazione (ad esempio, facendo ricorso alle categorie professionali e caricandole di questa responsabilità). Per la parte penale, invece, io credo che la scelta della depenalizzazione di molti reati sia una scelta congrua,

che obiettivamente crea una condizione di sovraffollamento insopportabile. Apprezzo la dichiarazione dello stato di emergenza e l'utilizzo di strumenti straordinari per la soluzione del problema delle carceri; ma accanto a questo, signor Ministro, la sollecito ad un intervento organizzativo e legislativo che modifichi profondamente il sistema che porta alla detenzione, riducendo i flussi in entrata nelle carceri e selezionando

debbono essere superate; quindi, nella sua scelta sull'edilizia carceraria, accanto allo sviluppo di nuovi padiglioni e di nuove carceri, la sollecito anche ad un'impostazione che diversifichi profondamente questo intervento del suo Dicastero. In questo ragionamento, credo che il Parlamento le sarà di grande utilità, perché i temi della riforma della giustizia, per la grandissima parte, trovano nelle Aule parlamentari la sede deputata alla definizione di questi procedimenti;

il clima che viene costruito in Parlamento dovrebbe basarsi su un confronto aperto alla ricerca di soluzioni che abbiano come obiettivo indiscusso la riqualificazione del sistema giudiziario, la riduzione dei tempi e l'eliminazione della farraginosità dei procedimenti, e quindi la certezza per il cittadino di avere questo servizio in termini qualificati ed efficaci, ma anche la certezza della pena e della sanzione. Non vi può infatti essere il dubbio che da un canto la scelta del Governo e della maggioranza sia quella di elevare la risposta punitiva dello Stato,

Paese, come lei ha già spiegato bene, e per assicurare a tutti i cittadini una risposta efficace e assolutamente equanime, allora credo che il Parlamento potrà essere un luogo eccellente in cui confrontarsi perché il Governo possa dispiegare la sua azione.

un'analisi che contiene anche quel dato sicuramente scioccante per i nostri cittadini dei 470 processi penali che ogni giorno vanno estinti per prescrizione e ciò ci fa davvero riflettere sull'efficienza di questo servizio. Abbiamo letto le sue proposte e i suoi obiettivi per il 2010, li condividiamo integralmente e ovviamente li abbiamo indicati come prioritari anche per questo ramo del Parlamento. Mi limiterò quindi solo a due brevi considerazioni. Innanzitutto vorrei

Lei prima ha citato il Governo Prodi, dicendo che in termini di giustizia è stato uno straordinario Governo delle buone intenzioni.

all'Esecutivo di cui peraltro era sottosegretario l'eruditissimo collega Li Gotti (plurilaureato, anche ad Oxford - anche se ha perso l'accento Harvard, come mi suggeriscono). In uno studio del Governo Prodi che si intitola: «Rapporto intermedio sulla revisione della spesa», redatto da una Commissione tecnica per la finanza pubblica presieduta dal professor Muraro dell'università di Padova,

«i principali risultati di questa comparazione rivelano come sia il livello della spesa pubblica in Italia» - per il settore giustizia - «sia il numero di magistrati per abitante non siano significativamente diversi da quelli degli altri Paesi europei pur evidenziando una durata media dei processi superiore a quella dei Paesi più avanzati». Questa è la considerazione che la Relazione motiva in maniera molto dettagliata, analizzando analizzando la spesa *pro capite* e il numero dei magistrati per ciascun Paese europeo, e dimostra come il problema italiano non sia legato alle risorse devolute al sistema giustizia, ma al loro utilizzo, alla disorganizzazione, all'approssimazione con la quale, purtroppo, esse vengono gestite; le risorse sono male organizzate, prevale la disorganizzazione. Come ha affermato il Ministro, non potrebbe essere diversamente, posto che ai vertici degli uffici giudiziari non ci sono *manager* in grado di far funzionare correttamente queste aziende di erogazione di un servizio quali sono i tribunali, ma ci sono giudici arrivati alla carriera dirigenziale solo per anzianità e che, per mentalità, sono anni luce lontani dalla capacità di gestire in maniera efficiente la loro struttura. Accantoniamo quindi l'affermazione, spesso ripetuta in maniera tralatizia, della mancanza di risorse nel settore giustizia, poiché le risorse ci sono e vanno bene organizzate. Aggiungo poi un passaggio sulla situazione assurda

siamo stati condannati a versare 118 milioni di euro per gli indennizzi legati alla legge Pinto. Prima si è parlato

della durata dei processi non ci sono precedenti in Europa. Invece, c'è un bellissimo articolo - ve lo consiglio, colleghi dell'opposizione - di Giovanna Ichino, pubblicato sulla rivista di Magistratura democratica (quindi non proprio una rivista di centrodestra), cui si cita l'esempio della Finlandia. Permettetemi di citarlo, in maniera che possa annotarlo anche il Ministro. In Finlandia, i tribunali e il Ministro della giustizia si accordano sulla negoziazione delle risorse da destinare ai tribunali sulla base dell'obbiettivo che i processi durino meno di un anno. In Finlandia le risorse vengono date dal Ministro della giustizia in maniera differenziata, a seconda dell'impegno del tribunale nella definizione in tempi ragionevoli dei processi. In Norvegia - ci spiega Giovanna Ichino - è stato raggiunto un accordo sulla durata delle procedure civili e penali da parte del Ministro della giustizia e del Parlamento.

la legge sul processo breve. Magari ci fosse la possibilità di negoziare direttamente le risorse fra il Ministro della giustizia e i distretti giudiziari, i tribunali, le corti d'appello! Purtroppo, questo Purtroppo, questo non è possibile. Assistiamo a una magistratura sindacalizzata, politicizzata, che si è arroccata e chiusa a riccio e che rifiuta qualsiasi proposta di riforma.

che divide la maggioranza dall'opposizione sul servizio giustizia e sui valori politici di riferimento nella riforma di questo servizio. Al Gruppo della Lega Nord, personalmente, la retorica vuota delle grandi riforme che poi non arrivano mai. A noi interessa un servizio giustizia adatto alle necessità del ventunesimo secolo e di un Paese europeo e moderno. Lei, signor Ministro, ha dimostrato di operare nella giusta direzione. Quindi, le auguriamo buon lavoro. Prosegua così. Signor Presidente, anche io vorrei augurare buon lavoro al Ministro, anche se la sua Relazione non ha assolutamente convinto né me né il Partito Democratico. Signor Ministro, lei è venuto a illustrare il suo programma sulla giustizia in un giorno particolarmente difficile. È un giorno in cui è stato consumato quello che noi abbiamo definito lo scempio della giustizia, perché proprio oggi in Senato è stato approvato da parte della maggioranza il disegno di legge sul processo breve.

Quando sono intervenuta nel dibattito, le ho chiesto se lei fosse davvero convinto che tutte le riforme che sono stato approvate o messe in campo in materia di giustizia e sicurezza, oltre che rispecchiare un progetto organico, fossero rispettose delle regole e dei valori della nostra Costituzione. Gliel'ho chiesto perché le norme che non rispondono alla Costituzione sono sono inefficaci. Lo dichiara con ritardo la Corte costituzionale. Il Paese perde un altro pezzo di giustizia e di rapidità della giustizia e, oltre tutto, l'operato della Corte costituzionale viene messo in discussione. Su queste premesse noi non possiamo certamente costruire un dialogo. Voglio anche dirle, signor Ministro, che sono profondamente colpita dal fatto che lei voglia condurre una forte lotta alla criminalità organizzata. Io sono convinta che tale intento sia estremamente utile e che debba essere condiviso. Se così è, però, signor Ministro, vuole spiegarmi per quale motivo, con il processo breve, voi avete azzerato la lotta contro la corruzione e contro i reati commessi dai pubblici amministratori?

la sfido - istituzionalmente - a presentare un disegno di legge che innalzi le pene per i reati in materia di corruzione e per i reati dei pubblici amministratori.

contemporaneamente al giudizio nei confronti degli amministratori corrotti sul piano contabile, il Governo e la maggioranza chiudono ogni possibilità di perseguire i reati contro la pubblica amministrazione. Ministro, di presentare un disegno di legge, su cui immediatamente noi daremo il nostro consenso. Voglio aggiungere che lei, tra l'altro, ha giustamente rivendicato di aver compiuto grandi passi in materia di rapporti internazionali. Signor Ministro, per conto del Ministero della giustizia sono stata due anni a Vienna ed ho stretto rapporti al fine di far approvare la Convenzione ONU sulla corruzione. Questa Convenzione è stata, tra l'altro, ratificata quest'anno con una legge di questo Governo e con essa noi ci siamo impegnati a rendere più efficace la lotta contro la corruzione

il nostro Stato non fa nulla per rendere più efficiente il processo, cioè non interviene sulla brevità con istituti e strumenti utili. Benissimo, facciamolo, perché siamo veramente stretti da un vincolo internazionale, e siamo intervenuti sul punto con una legge di ratifica dello Stato a tutto campo. Io le chiedo: ma lei che figura va a fare in sede internazionale se poi non rispetta questi impegni? PD).* Vorrei parlare poi della desertificazione delle procure (non credo di poter affrontare tutti gli argomenti che mi ero prefissa: lascerò pertanto il mio discorso Lei giustamente, signor Ministro, ha detto che avete raggiunto un accordo oggi alla Camera, dove è stato approvato un emendamento per cui coloro che saranno nominati uditori giudiziari nell'ultimo concorso andranno a riempire le sedi disagiate. quanto mi è stato riferito, non so se sia in questi termini, e me ne scuso, perché non ero alla Camera; ma se così è, signor Ministro, perché non possiamo fare una riforma che non sia semplicemente contingente ma a regime e che tenga conto oltretutto che tenga conto oltretutto anche dei valori cui non possiamo derogare? Quando il Consiglio superiore della magistratura, un organo di rilevanza costituzionale con cui lei non vuole dialogare, vi richiama

non rispecchia tali valori e quindi va corretto; su questo punto siamo disponibili a venirvi incontro i tutti modi, perché è nostro interesse che la giustizia funzioni. Voglio aggiungere anche che i politici e i magistrati di Reggio Calabria, da cui vi siete recati, vi hanno chiesto, tra l'altro, non solo di coprire le sedi e di mettere a loro disposizione magistrati e personale amministrativo ma ma anche di non abbassare la guardia contro la criminalità organizzata e quindi di non ridurre le misure che servono a contrastarla. Signor Ministro, lei ha rivendicato in questa sede il disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche:

La criminalità organizzata infatti si fonda anche su tutti quei reati satellitari, che però sono funzionali, sono la base di un sistema che consente alla stessa di proliferare e di riprodursi. Quindi, questa sua rivendicazione del disegno di legge, senza nessuna possibilità di apertura a modifiche, mi lascia sinceramente preoccupata. un'altra questione. Signor Ministro, lei ha dichiarato che il Consiglio superiore della magistratura sbaglia e che non c'è necessità di riforma delle circoscrizioni giudiziarie. Vorrei capire perché, signor Ministro; non mi è chiaro: soltanto perché lei è passato per alcuni uffici giudiziari e ha trovato che gli uffici di grandi dimensioni funzionano peggio di uffici di piccole dimensioni? mi sembra questa una risposta efficace ad un progetto che, invece, viene portato avanti da moltissimo tempo e che serve ad ottimizzare le risorse. Sul che i dirigenti degli uffici giudiziari debbano essere preparati, efficienti, all'altezza della situazione e che le buone pratiche debbano transitare da un ufficio all'altro e debbano essere seguite, siamo perfettamente d'accordo. Detto questo vorrei chiederle, signor Ministro, se rispetto alla Scuola superiore della magistratura stiamo andando avanti per la formazione dei magistrati. A questo punto, mi permetto di farle presente che, giustamente, il Consiglio superiore della magistratura ha raccomandato nel parere di considerare i rapporti tra i diversi organi dello Stato che hanno rilevanza costituzionale. Il fatto di esprimere, dopo il consenso per la nomina a dirigente dell'ufficio giudiziario, un ulteriore consenso sulla permanenza non rispecchia questi rapporti. Cambiamoli, per carità, con una modifica costituzionale ma, allo stato, questi poteri, Ministro, non ci sono. Allora, noi le chiediamo la riforma organica della giustizia civile, penale e amministrativa, una riforma della magistratura contabile e le chiediamo di intervenire in modo serio ed efficace nel mondo penitenziario, dove purtroppo i suicidi aumentano, e non mi pare che il piano carceri serva ad umanizzare il trattamento dei detenuti. Voglio aggiungere che appare molto pericolosa la previsione della detenzione domiciliare durante l'ultimo anno di pena, perché si tratta di un vero e proprio condono mascherato; su questo io richiamo la sua attenzione

dell'intervenuto processo breve, quindi agli imputati che andranno esenti da pena, anche i soggetti che, condannati anche per fatti di grave offensività e che magari sono recidivi, delinquenti abituali, potranno tornare a casa loro, in detenzione domiciliare, senza che le forze di polizia abbiano la possibilità di controllarli. Se questa è giustizia e sicurezza io le chiedo, signor Ministro,

a mo' di rimprovero, e a dir la verità ieri ci è stato anche ripetuto come un *refrain*, che il metro di indirizzo che deve guidare i provvedimenti in tema di giustizia è l'interesse dei cittadini. Allora, dopo aver ascoltato la sua Relazione, signor Ministro, e la sua replica, vorrei chiedere ai colleghi dell'opposizione, senza retorica e senza polemica: all'interesse di chi dovrebbero essere ascritte misure come quelle adottate o avviate finora? Nell'interesse di chi sono la riforma del processo civile e quella della professione forense, la riforma del processo penale e le misure di innovazione tecnologica e organizzativa, le norme antimafia e il pacchetto sicurezza? Nell'interesse di chi è una riforma del processo penale che garantisca effettiva parità tra accusa e difesa, o una norma che fissi i termini della ragionevole durata dei processi a fronte dei numeri che il Ministro ci ha illustrato e che dovrebbero far rabbrividire chiunque abbia a cuore la permanenza dell'Italia nel novero dei Paesi civili? Ancora: nell'interesse di chi va la risposta che il Governo ha messo in campo rispetto all'emergenza carceraria? Su quest'ultimo punto in particolare mi consenta di soffermarmi, signor Presidente. Perché a quanti si professano sempre attenti al principio dell'uguaglianza di fronte alla legge, nel quale tutti ci riconosciamo, non sfuggirà che vi è anche un'altra esigenza di civiltà, ed è l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla pena. La stessa pena, scontata oggi in due carceri differenti, magari anche poco distanti, può infatti assumere connotati completamente diversi. Anche tra una sezione e l'altra di uno stesso penitenziario può verificarsi il medesimo squilibrio: basti pensare all'esorbitante sproporzione di detenuti in attesa di giudizio, che dovrebbe indurre a qualche riflessione più profonda anche sull'uso della carcerazione preventiva. Lo abbiamo detto qui in occasione del dramma di Stefano Cucchi lo ripetiamo oggi: noi riteniamo che le istituzioni siano tanto più credibili quanto più riescono a fare luce al proprio interno sui problemi e sulle responsabilità individuali. Allo stesso tempo, però, sarebbe auspicabile intraprendere una riflessione a tutto campo ed evitare inutili demagogie. Senatore Li Gotti, io non ho mai creduto che l'ignoranza fosse un peccato. Anzi, è probabilmente il presupposto della libertà, perché se sapessimo tutto i nostri comportamenti sarebbero obbligati. lei, per essere stato in quest'Aula, dovrebbe sapere che un piano carceri poteva essere scritto solo dopo che un capitolo apposito fosse stato stanziato nell'ultima finanziaria. Le consiglio di andare a consultare quel testo.

i diritti dei detenuti ed i diritti degli uomini dello Stato che ogni giorno si occupano di loro. Per ricordare, senatrice Della Monica, accanto all'allarmante bollettino dei suicidi in carcere, che preoccupa anche noi, un altro bollettino: quello sei volte più grande dei detenuti che ogni anno tentano di togliersi la vita e vengono salvati dagli agenti di Polizia penitenziaria, che rappresentano l'altra faccia della luna di cui troppo spesso ci si dimentica. Per ammettere che anche le migliori intenzioni dei paladini dei diritti umani ogni tanto si scontrano con le piccole ipocrisie quotidiane. Basti pensare al carcere di Pisa.

Ebbene noi, signor Presidente, crediamo nella forza delle istituzioni, nella presenza dello Stato e nella cooperazione fra chi, a vario titolo, se ne fa interprete: nel Governo, nel Parlamento, con chi con chi indossa una divisa e chi ha la toga sulle spalle. Ed è bene in tal senso che non si perda occasione per rivendicare con orgoglio quale cappio mortale sia stato stretto in questa legislatura intorno al collo della mafia, grazie all'iniziativa politica del Governo e della maggioranza *(Applausi dimostrata nei confronti degli apparati dello Stato. Perché, signor Presidente, onorevole Ministro, lo Stato è uno solo, e noi non ci faremo mai incantare dalla falsa coscienza di chi vorrebbe reintrodurre sotto mentite spoglie il paradigma del doppio Stato, contrapponendo ad ogni arresto di latitante, ad ogni arresto eccellente, i magistrati buoni e il Governo cattivo. *(Applausi dal suscitato notevole rammarico, tanto che il comunicato di oggi suona come parziale ricompensa, le polemica inscenate nei giorni scorsi dall'Associazione nazionale magistrati contro il tentativo del Governo di far fronte alle carenze di organico nelle sedi disagiate, che sono anche le sedi più esposte. Perché se la lotta alla criminalità organizzata è una priorità per tutti, essa si nutre del sacrificio e della buona volontà di tutti, e non si dà al Paese un bello spettacolo di sé minacciando di infrangere la solidarietà istituzionale in nome di una visione corporativa. Signor Presidente, noi ci auguriamo che la stagione del pregiudizio, del "no" a prescindere a qualsiasi tentativo di modernizzazione, abbia presto fine. Anche perché la sfida che ci aspetta, e che lei, Ministro, ci ha ricordato, è ambiziosa e non consente veti preventivi. Mi riferisco alla riforma costituzionale della giustizia: la prima e più importante delle riforme istituzionali, per garantire ai cittadini un sistema più equo, al Paese una maggiore competitività, e consentire a quella maggioranza silenziosa di magistrati che ogni giorno compie il proprio dovere di recuperare presso il popolo italiano la fiducia in parte smarrita a causa di una minoranza rumorosa di toghe che all'idea della prestazione di un servizio ha preferito l'idea dell'esercizio di un potere, anche a fini impropri.

che, come lei ci ha detto signor Ministro, sia ricondotto al suo spirito originario, mondato dalle bramosie di assurgere a ruoli che non gli sono propri e libero dalla morsa della spartizione correntizia. sovranità del popolo, ricucendo un equilibrio spezzato e disinnescando una volta per tutte un conflitto che da quindici anni avvelena i pozzi della nostra democrazia. Qualsiasi sia la strada che si deciderà di percorrere, non si tratterà soltanto di porre fine alla persecuzione giudiziaria nei confronti di un Presidente del Consiglio *hic et nunc*, ma di ripristinare i pesi e contrappesi di un sistema ormai sbilanciato al punto da porre in dubbio l'origine stessa della sovranità. È questo l'auspicio di quanti avrebbero voluto che la riflessione del centrodestra sulla candidatura in Campania si svolgesse solo intorno a considerazioni politiche, e non alle accuse di qualche pentito risalenti al secolo scorso e sfornate a rate con singolare "puntualità". Di quanti avrebbero preferito che alle primarie in Puglia partecipassero soltanto gli elettori del centrosinistra, e non il fantasma di un avviso di garanzia tempestivamente notificato a mezzo stampa alla vigilia della consultazione. Credo che in fondo questo sia anche l'auspicio dei colleghi dell'UDC, che in questi giorni hanno sentito sulla pelle di Calogero Mannino le piaghe di un calvario lungo quasi due decenni, anche se talvolta sembrano stentare a trarne le conseguenze. Certamente è l'auspicio di chi ritiene che fra le funzioni della magistratura non vi possa essere quella di decidere della composizione delle istituzioni che rappresentano il popolo sovrano. E di coloro che, appena un mese fa, in piazza Duomo a Milano, hanno saputo scorgere le conseguenze di campagne d'odio che si alimentano dell'uso politico della giustizia, e anche della gestione impropria di sedicenti pentiti sulla quale spero che in un giorno non lontano, in Parlamento, saremo chiamati a fare luce per mettere fine ad una stagione non edificante per l'Italia.

Grazie perché, in fase di replica, il ministro Alfano ha voluto ricordare gli impegni presi a seguito delle proposte dei radicali. Spero che dalle parole si passi ai fatti e anche che, in sede di dibattito presso le Nazioni Unite il 7 febbraio prossimo, quando il Consiglio delle Nazioni Unite sui diritti umani parlerà dell'Italia, si voglia denunciare non la crisi della giustizia italiana, ma il collasso della giustizia italiana. Mi asterrò anche sulla mozione dell'Italia dei Valori da cui mi separano i valori relativamente all'amministrazione della giustizia.

ha ricordato gli impegni presi sulla base di documenti scritti anche dai radicali, impegni che però purtroppo sono rimasti tali e non si sono trasformati in atti di Governo e neanche in atti parlamentari. Nella replica, signor Ministro, lei ha detto che la strada scelta dal Governo non è quella di un'altra amnistia e di un altro indulto, ma le chiedo: e le 200.000 prescrizioni di ogni anno cosa sono se non un'amnistia di classe,

che il legislatore facesse quello che è il suo compito, ossia fare le leggi nell'interesse dei cittadini italiani. Bene, oggi Francesco Zanardi è al diciassettesimo giorno di sciopero della fame. Le risposte, purtroppo, non sono state Il 4 gennaio, in Piazza Montecitorio, Francesco e Manuel si sono rivolti ai Presidenti del Parlamento e delle Commissioni parlamentari giustizia di Camera e Senato per chiedere la calendarizzazione delle proposte di legge depositate dai diversi Gruppi politici sulle unioni civili e sul matrimonio gay. Io ero presente a quell'iniziativa anche con l'associazione radicale "Certi diritti". Mancavano tanti parlamentari, ma soprattutto è mancata una risposta del Parlamento per i tanti Francesco e Manuel, per le tante coppie che chiedono diritti

a chiedere la calendarizzazione, l'impegno da parte della Commissione giustizia a riprendere un dibattito su temi che stanno a cuore a tanti cittadini che hanno la sfortuna di volersi bene, ma di appartenere allo stesso sesso.

Signor Presidente, oggi il senatore Li Gotti, con quel suo tratto elegante che ha mutuato solo in parte dal capo del suo partito che, per eleganza, non può prendere ovviamente lezioni da nessuno avendo toccato dei vertici inarrivabili, ha detto a noi della maggioranza,

Ora, mi sono fermato a considerarmi e mi sono anche riconosciuto. Certo, sono un somaro in diritto penale e in procedura penale; ma ho avuto un grande conforto, perché se il senatore Li Gotti ha ritenuto di dire con tanta forza che siamo dei somari, evidentemente deve avere una forza in sé e una consapevolezza dell'io che lo fa grande ai miei occhi.